la scorsa settimana si è svolto in quest'Aula è svolto in quest'Aula un dibattito molto approfondito, alla presenza del ministro Padoa-Schioppa, c'è stato un confronto e, in alcuni casi, anche uno scontro; i giornali hanno scritto addirittura che in alcuni casi si era superato il limite di guardia. Questa mattina ci doveva essere Questa mattina ci doveva essere l'insediamento del generale D'Arrigo al comando della Guardia di finanza e, dalle agenzie, apprendiamo che è stato rinviato. C'è addirittura un'agenzia che riferisce del picchetto d'onore già schierato, mentre poi l'insediamento non si è tenuto. So che questa mattina questo problema era già stato sollevato,

Vi prego di prendere posto. C'è un grande fastidio rilevato dai colleghi che stanno ascoltando. MATTEOLI

Si è cacciato il generale Speciale e si è sostenuto in quest'Aula che c'era il diritto da parte del del Governo di cacciarlo, ma credo che da parte del Governo ci sia anche il dovere di insediare il nuovo Comandante generale della Guardia di finanza. Da una parte, è stata cacciata una persona, dall'altra non si è stati in condizione di insediarne un'altra. La Guardia di finanza sta vivendo un momento di grande confusione. Credo sia opportuno che il Governo venga a riferire su quanto è accaduto questa mattina e soprattutto venga a chiarire quando e come sarà insediato il nuovo Comandante generale della Guardia di finanza. Non possiamo leggere sulle agenzie che molto probabilmente domani mattina la Corte dei conti registrerà il decreto. Non è possibile che siano le agenzie a dettare il calendario del Governo in relazione alla Guardia di finanza. Si riferisca nell'Aula del Senato cosa è avvenuto questa mattina e perché non si è insediato il nuovo Comandante generale della Guardia di finanza.

il Presidente della Repubblica possa avere mandato un messaggio che, secondo quanto è contenuto nelle indiscrezioni delle agenzie, sollecita l'approvazione di un provvedimento, prendendo evidentemente parte, visto che di fatto indica che la riforma che è stata varata dal Parlamento (non dico da quale parte, ma dal Parlamento) nella scorsa legislatura, in piena legittimità democratica, deve essere abrogata.

non ha alcuna considerazione nei nostri confronti e divulga intercettazioni di ogni tipo, calpestando l'articolo 68 della Costituzione. Adesso c'è anche il Capo dello Stato che ci dice quali leggi dobbiamo approvare e quali no. Ma c'è qualcuno in questo Parlamento che ha la schiena dritta e vuole rivendicare il fatto che siamo noi gli eletti dal popolo e siamo soltanto noi che possiamo decidere cosa fare e cosa non fare, quali leggi approvare e quali non approvare?

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Matteoli, ricordo che questa mattina più di un senatore

Sono convinto che, poiché i lavori del Senato sono pubblici, le preoccupazioni espresse in quest'Aula siano state recepite da chi rappresentava il Governo qui e fuori quell'avvenimento che a partire dal senatore Pastore sembrava si dovesse verificare, non si è verificato. Raccolgo, in ogni caso, la sua raccomandazione di prendere contatti con il Governo per vedere se si riesce ad ottenere in un dibattito un chiarimento sul punto. Per quanto riguarda poi l'intervento del senatore Castelli, il Presidente della Repubblica, secondo me, non ha fatto altro che esprimere in una lettera privata una sua preoccupazione che non tocca minimamente il merito:

ha inviato un messaggio alle Camere, la Commissione può discutere entrando nel merito delle questioni. Tutto qui. Ritengo che aprire una discussione su questo punto sia assolutamente sbagliato, non possibile e, comunque, inaccettabile.

e quindi non pensavo di intervenire sul punto, perché mai avrei potuto immaginare che il Presidente della Repubblica avesse potuto inviarle una lettera come quella che le ha inviato. Mi dispiace anche per il senatore Salvi, che ha mostrato una grande indignazione sul punto, addirittura arrivando a chiedere la censura del senatore Castelli. Probabilmente è vero che nei sessant'anni precedenti non vi è mai stato in queste Aule un intervento come quello del senatore Castelli, ma probabilmente è anche vero che nei sessant'anni precedenti non vi è stata una lettera come quella che il Presidente della Repubblica le ha inviato. Signor Presidente, vorrei dire però una cosa; mi scusi, ma il problema è importante: lei ha parlato di una lettera privata, che poi tanto privata non doveva essere perché è stata correttamente - come lei ha ritenuto di dover fare - trasmessa al Presidente della Commissione giustizia. Ma veda, signor Presidente, il problema non è la preoccupazione del Capo dello Stato di rendere più veloci i lavori del Senato o della Camera in termini generali; nel caso di specie, signor Presidente, come ella ci ha ricordato poc'anzi,

Non intendo aprire una discussione, mi avvio a concludere. Dal mio punto di vista, le dico con molta tranquillità che considero l'intervento del Presidente della Repubblica un intervento effettuato al di fuori delle competenze che gli sono assegnate dalla Costituzione.

propongo di sviluppare oggi il dibattito generale sul punto che è stato discusso questa mattina, cioè la sicurezza sui luoghi di lavoro. portiamo avanti e concludiamo la discussione generale, se abbiamo tempo anche le repliche del relatore e del Governo. Domani mattina, in ogni caso, verrà aperta la discussione

colleghe senatrici e onorevoli colleghi senatori, ripeto le cifre che già sono state riferite questa mattina all'inizio del dibattito. Sono cifre imponenti, importanti e ci danno la misura di quanto la situazione sia drammatica. 1.300 morti, più di un milione di infortuni ufficiali che colpiscono maggiormente lavoratori immigrati e donne, maggiormente le classi d'età più avanzate: per chi pensa che si debba allungare l'età pensionabile, questo è un dato molto interessante. Ci sono più infortuni presso le classi e le età successive ai quarant'anni, stando ai dati INAIL. A tali cifre vanno aggiunti i circa 200.000 infortuni non denunciati a causa del lavoro nero e l'insorgenza di numerose patologie che coinvolgono uomini e donne per via della loro attività di lavoro, scarsamente denunciate all'INAIL e ancora più scarsamente riconosciute. L'Organizzazione internazionale del lavoro ritiene che in Europa le morti per malattie di origine professionale siano il quadruplo di quelle per infortuni. Di questo scandalo e di questo conflitto tra capitale e lavoro ci stiamo occupando con il provvedimento in esame; credo che stiamo facendo la cosa giusta ed è - se mi è permesso - mi è permesso - una cosa giusta di sinistra, una di quelle che la gente e il popolo che ci ha votato aspetta. Non è sufficiente una nuova normativa per la salute e la sicurezza del lavoro, ma bisogna intervenire anche sugli aspetti che concorrono a determinare il peggioramento delle condizioni del lavoro: prioritariamente sul tema della precarietà del lavoro, come ci dicono con chiarezza i dati INAIL, nella lotta contro il lavoro nero irregolare e sommerso. tutela della salute nei luoghi di lavoro si intende il tema più generale della salute intesa in senso ampio. I determinanti della salute sono i fattori che condizionano il peso delle malattie nella società e influiscono in modo significativo sulla salute della popolazione. Solitamente essi sono raggruppati in categorie quali il comportamento personale e lo stile di vita, i fattori sociali, che possono essere vantaggiosi o svantaggiosi, condizioni di vita e di lavoro, l'accesso ai servizi. I fattori socioeconomici e gli stili di vita condizionano la salute al 40-50 per cento; lo stato e le condizioni dell'ambiente per il 20-30 per cento; l'eredità genetica e i servizi sanitari solo per il 10-15 Lo stile di vita, quindi, è fortemente influenzato da altri determinanti, fra cui l'occupazione, il reddito, l'istruzione e la cultura. Questi elementi influiscono sullo stile di vita dei singoli individui. A sua volta, la condizione socioeconomica costituisce un importante determinante dello stato di salute. Tendenzialmente le persone meno abbienti, meno istruite, che svolgono un lavoro più rischioso, più pesante e faticoso si ammalano di più e muoiono di più. Il miglioramento della salute e la riduzione delle disuguaglianze nella salute è un obiettivo in sé e costituisce una condizione rilevante dello sviluppo economico. Si pensi, sempre stando ai dati INAIL, a quei tre punti di PIL in meno, oltre al costo umano derivato da infortuni e malattie professionali. pertanto su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non solo afferma un diritto, quello ad ottenere il migliore livello di salute ottenibile, come sottolinea l'Organizzazione mondiale della sanità, ma incide direttamente sulla disuguaglianza sociale. Per questo, intervenendo su tale tema, così come si è fatto nell'ultimo anno con vari provvedimenti (penso al decreto Bersani, alle norme importanti contenute nella legge finanziaria, al disegno di legge che abbiamo votato solo ieri sul grave sfruttamento dei lavoratori irregolari), stiamo assumendo una misura che certo migliora la condizione del lavoro, ma migliora anche complessivamente la condizione di disuguaglianza di questo Paese. In tale ottica va concepita questa misura, così come in tale ottica i luoghi di lavoro devono essere non solo sicuri

Del resto, l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo 41 della Costituzione pone limiti all'iniziativa economica privata là dove parla di utilità sociale e di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità della persona. Lo Statuto dei lavoratori, all'articolo 9, sancisce il diritto dei lavoratori a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Proprio dal protagonismo del movimento operaio, del movimento delle donne e dei movimenti sociali, la centralità della salute è diventata la base per affermare la propria soggettività, i diritti, la cittadinanza piena. Da tali movimenti prende vita una storia che viene da lontano, che ha segnato il mondo del lavoro punteggiato punteggiato di tragedie, che voglio citare per la loro emblematicità. Ce ne sono tante: ne ricordo solo alcune, quelle che confusamente ci vengono in mente immediatamente. Ricordo Marcinelle, perché fu una strage enorme, ma soprattutto perché in quel caso gli immigrati eravamo noi, perché parla di questa doppia condizione che a volte sembriamo aver dimenticato. Penso a Seveso, perché quello è un punto che segna un drammatico rapporto tra ambiente di lavoro-produzione del lavoro e invasione devastante dell'ambiente circostante. Penso a Porto Marghera, che tanti lutti addusse a tutto il movimento e ai lavoratori di quella fabbrica. E soprattutto penso alla lotta per la messa al bando dell'amianto.

Oggi, come allora, il tema della partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso la contrattazione collettiva, con i loro delegati sindacali, le RSU o le RSA, con gli RLS (cioè i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), per la sicurezza), è la condizione per un'applicazione viva, dialettica della legge e per una ricomposizione di qualità del lavoro e dell'ambiente, da un lato, e per politiche industriali e produttive, dall'altro. Il nostro Paese è quello con il mercato del lavoro più flessibile d'Europa e noi sappiamo che salute e sicurezza del lavoro dipendono da elementi molteplici, dalla disarticolazione produttiva derivante dalle numerose esternalizzazioni e dalla filiera di appalti e subappalti; dipendono dalla precarietà del lavoro; dipendono dalla particolarità del lavoro autonomo, spesso lavoro subordinato mascherato; dipendono, ancora, da illegalità e criminalità organizzata, ma anche da un'insufficiente applicazione dei princìpi della prevenzione, dai ritardi, dall'indifferenza nell'assunzione della specificità delle lavoratrici e della dimensione di genere oltre ai rischi diretti legati a gravidanze e allattamento. Evidente è il legame tra aumento degli infortuni e flessibilità del lavoro, perché l'abbattimento dei costi del lavoro si è ottenuto con l'introduzione di nuove tipologie di lavoro, moltiplicando precarietà, ricattabilità dei lavoratori, imposizione di ritmi più intensi, ma anche considerando la sicurezza come un costo da tagliare. Non a caso, i tassi di infortunio sono più alti tra i lavoratori precari, tra gli immigrati, così come sono in crescita gli infortuni anche con esito mortale tra le donne. Nel

Ma è necessario e urgente un intervento complessivo e articolato per combattere il lavoro nero, irregolare e sommerso, il lavoro minorile, quello in nero degli immigrati, per superare la legge n. 30 del 2003 e la precarietà, per gli ammortizzatori sociali, per la democrazia nei luoghi di lavoro: questi sono, seppure non direttamente, agenti di sicurezza e salute del lavoro, costruiscono un contesto dentro il quale una politica di sicurezza può crescere e ampliarsi. Devo sottolineare - questa mattina è già stato fatto dal senatore Zuccherini

quegli arricchimenti del testo di legge che facevano riferimento alla specificità del lavoro delle donne e alla necessità di pensare in termini di prevenzione, di valutazione dei rischi e di misure da intraprendere anche in termini di genere. Quello che manca, purtroppo, invece è un intervento preciso sul lavoro domestico che, come è stato detto, è foriero di una quantità di incidenti che si svolgono dentro le mura domestiche, nella piena solitudine di chi lavora. È un provvedimento che riteniamo urgente, sul quale dobbiamo lavorare e sul quale penso che la Commissione dovrà spendere parte del suo tempo perché possa essere introdotto in questo testo. Ho già detto che in questo anno possiamo essere, in qualche modo, se non soddisfatti, per lo meno

di intervento nel mondo del lavoro: penso all'introduzione degli indici di congruità, all'estensione della dichiarazione unica di regolarità contributiva, ma non li voglio citare tutti. C'è un punto di concretezza: questi obiettivi vanno concretamente perseguiti, non possono soltanto essere enunciati. Quindi, bisogna pensare alle difficoltà economiche che si stanno incontrando nel previsto rafforzamento della capacità ispettiva, da ottenersi mediante il potenziamento di 60 unità dell'organico del Comando dei carabinieri; ma bisogna pensare anche all'incremento fino a 300 unità del numero di ispettori del lavoro.

A tal proposito, non è stato certo piacevole ascoltare in Commissione lavoro e poi leggere dalle colonne di qualche giornale che sarebbero già terminati i soldi a tanto destinati: si rischia davvero di dare uno spettacolo

questa situazione, insieme a quella dell'irregolarità, che genera fragilità, precarietà, ricattabilità, venga affrontata. Occorre, infine, che il Senato si attivi, da un lato, per ratificare la Convenzione ONU sui diritti dei migranti, dall'altro lato, perché le aziende italiane che operano all'estero, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, applichino la legge italiana, quando questa sia migliore di quella del Paese in cui l'azienda opera. Anche così renderemo un buon servizio ai lavoratori e al diritto. Poiché prima ho citato Medicina Democratica

in massimo grado la concentrazione della nocività e la spoliazione della salute, ma era anche il luogo dove il movimento operaio aveva chiarito a sé e agli altri che la lotta collettiva per la salute collettiva investiva tutto il modo di produzione e lo contestava in ciò di cui era più geloso: la sua falsa razionalità».

Mi scusi, lei ha chiesto di far intervenire prima il senatore Amato: a che titolo lo chiede, scusi?

*(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge delega oggi in discussione è stata ottimamente rappresentata dal senatore Carrara e dagli altri colleghi fin qui intervenuti. Mi limiterò, pertanto, ad esprimere alcune considerazioni relative a taluni punti critici del testo in esame. Vorrei partire subito dalla sottolineatura di un principio che, a me, non pare pienamente recepito nel disegno di legge delega. Ritengo infatti che ogni provvedimento di legge a carattere sociale, nello stabilire le proprie finalità, dovrebbe sempre e comunque tenere in considerazione la funzione sociale dell'impresa. Funzione sociale che consiste nel creare profitto e ricchezza secondo la logica del mercato e non nel caricarsi di obblighi formali e nel sostituirsi ad enti previdenziali o, peggio, ad autorità che non riescono a controllare l'applicazione di regole giustamente emanate a tutela dei lavoratori e della loro salute. Lo dico perché, leggendo l'articolo 4 del testo proposto dalla 11a Commissione, ad integrazione dell'articolato presentato dal Governo, non ho trovato questa considerazione per il ruolo ed il valore sociale dell'impresa. A colpirmi negativamente e a preoccuparmi politicamente, non sono soltanto la tipologia e la quantità di sanzioni previste per l'impresa, ma è anche, e soprattutto, la filosofia che ispira tale foga sanzionatoria. infatti non può essere caricata di ogni responsabilità, senza peraltro distinzioni di sorta in ordine alle dimensioni aziendali, e senza un forte richiamo alla responsabilità di chi ha il compito istituzionale di prevenire e di controllare, a livello nazionale, come a livello locale. livello locale. La complessa situazione che sta dietro questo provvedimento potrebbe, in realtà, essere letta semplicemente, cioè nel seguente modo: c'è un Governo che, non essendo riuscito ad organizzare in modo efficiente la rete dei pubblici poteri adibiti alla prevenzione e ai controlli, ha deciso di riversare, di fatto, sull'impresa gli oneri e le responsabilità dell'inefficienza della macchina statale.

Peraltro, esaminando i dati in nostro possesso, risulta che la maggior parte degli incidenti sul lavoro non avviene in ambito aziendale. Vi faccio un esempio concreto. La mia Regione di appartenenza, la rossa Toscana, detiene purtroppo, con poche altre, il triste primato degli infortuni sul lavoro, tanto che dal 1° gennaio al 22 maggio 2007 sono stati registrati 39 infortuni mortali. nella relazione presentata il 29 maggio 2007 dalla direzione dell'ispettorato regionale del lavoro alla speciale commissione del Consiglio regionale della Toscana, non solo è stato dimostrato che gli infortuni sul lavoro non sono in crescita, neppure nel delicato settore dell'edilizia, ma è stato anche precisato che, dei suddetti 39 incidenti, otto non sono stati riconosciuti dall'INAIL come infortuni sul lavoro, uno è stato semplicemente considerato un malore sul luogo di lavoro, tre sono avvenuti per cadute dall'alto e sei per schiacciamento o investimento, mentre ben 21 si sono si sono verificati sulla strada, ripeto, sulla strada! Ecco, è dalla realtà delle cifre che bisognerebbe forse partire, onde evitare il condizionamento di visioni o di affermazioni ideologiche. Resta, infine, il fatto che, da un disegno di legge che delega al Governo l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, mi sarei aspettato un maggior coinvolgimento delle Regioni e una più stringente sottolineatura della collaborazione che, in questo campo, deve necessariamente sussistere tra amministrazioni decentrate e Governo centrale. Lo dico anche perché non sempre le Regioni mettono in cantiere risorse ed iniziative atte a contrastare efficacemente, sul piano locale, gli incidenti sul lavoro o le violazioni alle norme di sicurezza. La mia Regione, ad esempio, nel bilancio di previsione 2007 ha ridotto il finanziamento previsto dal programma regionale di sviluppo per la qualità e la sicurezza del lavoro, scendendo da 8,5 a 5 milioni di euro. Un taglio Un taglio consistente, che lascia sconcertati, specie a fronte di tanti discorsi retorici sulle cosiddette morti bianche e di tante, troppe, spese inutili, largamente finanziate dal bilancio regionale. Credo, insomma, che sia doveroso trovare il modo di coniugare solidarietà e sviluppo, tutelando i lavoratori e il loro diritto alla salute, ma rispettando anche l'impresa, senza la quale non può esservi il lavoro e il conseguente diritto alla salute che su di esso si fonda. Per far questo occorre però recuperare, sul piano concettuale prima ancora che politico, il senso della realtà e della misura. Non mi pare che il disegno di legge oggi in discussione vada in questa direzione. Peccato, perché è un'occasione persa. Un'occasione persa, la cui responsabilità politica è tutta dei proponenti.

che si possa segnare oggi una pagina di speranza, per quei milioni di lavoratori che quotidianamente, con la loro fatica, portano avanti il Paese e lo fanno crescere.

negli ultimi anni quella Regione, quella stessa che produce una così larga parte della ricchezza nazionale, svetta nella triste classifica delle morti bianche e degli infortuni. Secondo le statistiche ufficiali, solo nel 2005 sono stati ben 2.354 gli infortuni mortali o ad elevata gravità verificatisi in Italia. Nello specifico, sono deceduti 1.482 lavoratori, mentre 872 sono rimasti permanentemente invalidi in maniera particolarmente grave. Di questi infortuni 444 sono avvenuti in Lombardia, quasi il 20 per cento, e il 60 per cento degli infortuni gravi o mortali si concentra nel Nord Italia. E questa è la fotografia ufficiale. Poi ce n'è un'altra, rappresentata da quei lavoratori, non solo immigrati, che non sono registrati come tali e da quei lavoratori che sono rimasti vittime di incidenti stradali perché stanchi e affaticati dal lavoro precedente. E muoiono anche altri lavoratori, vittime di esposizione ad agenti cancerogeni e tossici, per i quali quasi mai o a grande fatica si riesce a dimostrare che la causa della morte è il lavoro. Ogni giorno si compie una strage per il lavoro, tanto più grave quanto più culturalmente accettata. E questo avviene in un contesto in cui gli infortuni sul lavoro, tra tutte le tipologie e i settori, sono più di 900.000 all'anno. Questi numeri aiutano a capire. Aiutano a capire che morire di lavoro non è una cosa scontata o inevitabile: un quarto delle morti bianche avviene per caduta dall'alto, il 15 per cento per la caduta di oggetti. Sarebbe bastato un casco o una imbracatura per salvare delle vite, ma in quei cantieri i caschi non c'erano e forse qualcuno aveva pensato che le imbracature avrebbero rallentato il lavoro. cento degli infortunati ha meno di 35 anni. Trovare il motivo di ciò non è difficile. Sono infatti i più giovani ad essere esposti a lavori precari che, per la loro stessa natura, sono caratterizzati da un livello di sicurezza nettamente inferiore alla media. Perché mai un datore di lavoro dovrebbe investire sulla sicurezza di qualcuno che, al più, lavorerà per lui per 4 mesi? Troppo spesso un padroncino pensa che un lavoratore temporaneo non sia un patrimonio per l'azienda e, pertanto, non sia economicamente sensato investire su di lui. Tutto questo è tristemente confermato dai dati INAIL. I lavoratori interinali, infatti, sono in maggioranza uomini con meno di 40 anni e un basso livello di istruzione. Un quarto di questi sono lavoratori extracomunitari principalmente impiegati in lavori stagionali con forte caratterizzazione manuale: manifattura, edilizia e agricoltura. Nel caso degli infortuni per lavoratori temporanei, ben il 75 per cento si verifica nel Nord del Paese, a causa del massiccio utilizzo di tipologie di contratto flessibile in Lombardia ed Emilia Romagna. Gli effetti perversi della precarizzazione del lavoro, come emerge crudamente dai numeri, non riguardano solo l'accesso ai diritti sociali, ma anche lo stesso diritto alla vita. È per questo che dobbiamo esprimere oggi soddisfazione per il lavoro celere svolto in Commissione. Il provvedimento, presentato dal Governo ad aprile, è ora in Aula e siamo certi che la Camera sentirà, come del resto sta avvenendo in Senato, l'urgenza di questo impegno. Servono norme più forti e nette. Non vi possono essere rinunce al valore della scelta di prevedere, insieme a un'ampia delega in grado di affrontare il complesso delle norme, alcuni interventi puntuali e di immediata attuazione. Tutto questo rafforza il percorso che le istituzioni devono fare per mettere la parola fine all'inaccettabile situazione di cui ho detto prima. Certamente queste norme sono solo una parte della soluzione: la forte diffusione del lavoro nero contribuisce in modo decisivo ad aumentare la rischiosità dei luoghi di lavoro; buona parte delle morti bianche, infatti, riguarda lavoratori assunti in nero, spesso anche immigrati, senza tutela alcuna. Nell'edilizia un lavoratore su sei che muore è un migrante. Le soluzioni a questi problemi sono a portata di mano: servono investimenti in sicurezza, formazione ed informazione. Ciò nonostante, la ricerca esasperata del profitto, il desiderio malato e miope del contenimento dei costi, la scarsa legalità che caratterizza vaste aree dell'Italia si ergono a barriera contro una cultura del lavoro sicuro. L'ignoranza dei diritti e delle norme è senza dubbio una componente fondamentale di tutto questo. Infortuni e morti non costituiscono solo una situazione umanamente intollerabile, ma anche economicamente insensata, dati gli alti costi che ricadono sulla società. «E' assurdo che si debba morire sul lavoro. Abbiamo il dovere istituzionale di reagire, di indignarci, di gettare l'allarme, di sollecitare risposte». Queste dure parole del Presidente della Repubblica, questo monito, oggi hanno una prima, positiva, risposta. Speriamo che un clima coeso delle istituzioni rafforzi e acceleri l'azione di tutti, tanto delle Camere quanto del Governo. Morire sul lavoro non è un fatto ineluttabile, è un fatto inaccettabile. La restituzione al Paese della sua dignità passa oggi attraverso una scelta netta: cancellare dalla nostra storia questa traccia di sangue che ha macchiato l'Italia.

nei confronti di questo testo e alcuni suggerimenti che, in parte, sono presenti sotto forma di emendamenti, proprio perché il testo unico possa recepire le direttive comunitarie senza intaccare, come nei desideri del Governo di fatto non perfettamente realizzati, l'equilibrio tra lo Stato e le Regioni e per mantenere quanto più uniforme nel territorio questo intervento. Quindi, ripeto, è condivisibile in assoluto lo sforzo di riordinare, coordinare, armonizzare, semplificare le disposizioni di legge, e credo che il centro-destra su questo non possa che essere d'accordissimo, dal momento che l'ha portato sempre avanti come

Ed ecco perché sento il dovere di intervenire segnalando alcune defezioni in questa legge. Per esempio, non c'è un vero e proprio declarato, chiaro coordinamento tra i provvedimenti che investono la molteplicità delle deleghe dei vari Ministri; cioè permane ancora, in questo testo, una certa confusione circa gli interventi dei vari Ministeri. Addirittura, anche la collegialità dell'intervento tra i vari organi ministeriali in parte viene enunciata ed auspicata ma, di fatto, non viene chiarita.

soprattutto in materia di monitoraggio, controllo della verifica, modalità dell'organizzazione del sistema di partecipazione e concertazione. Sì, è vero,

al ruolo delle Agenzie, della Conferenza delle Regioni, delle società scientifiche. Non credo, quindi, che in una legge non ci debba essere già un'indicazione che dia un atto di indirizzo alle linee guida che, come sappiamo, troppo spesso vengono riservate soltanto ai tecnici che - ahimé sono gli stessi che oggi necessitano di questa legge perché nelle precedenti hanno lasciato delle defezioni. Spero che ne abbiano fatto tesoro; comunque ribadisco che un Parlamento debba dare questi criteri.

che ciò è dovuto alle proprie ideologie politiche e non alla realtà del Paese perché veramente è assurdo pensare che esistano ancora quelle realtà che sono state enunciate. Ce ne sono di sicuro di peggiori e su quelle dobbiamo intervenire, però, non cerchiamo di tracciare un'immagine che non ha Un'altra critica riguarda il mancato recepimento di alcune importanti direttive europee riguardanti l'amianto, il rumore e gli agenti fisici (per esempio le vibrazioni).

E ancora: vogliamo intervenire, una volta per sempre, sul lavoro flessibile? O volete annullarlo per sempre e pensare che non sia servito a niente? Andatelo a dire alle decine di migliaia di giovani e meno giovani, soprattutto quei meno giovani che purtroppo, per una serie di cause, hanno dovuto abbandonare il proprio lavoro e solo con il lavoro flessibile sono riusciti a raggiungere il numero di anni necessario per poter avere la pensione. Non so se questa carenza di intervento sul lavoro flessibile è legata ad un indirizzo

dovremmo essere un po' più pignoli nell'indicare cosa sia la buona tecnica e cosa la prassi. Infatti, la buona tecnica in genere è molto precisa, ma qui nel testo unico non è specificata. La prassi è legata a comportamenti condivisi che non sempre sono i comportamenti più adatti; quindi, rimanere nel generico vuol dire cadere negli errori del passato e di fatto avere una legge che ancora non

la posizione della Commissione sanità, che peraltro non è pervenuta; infatti, è stata letta dopo e me ne dispiace. Spero venga recepita, perché ancora una volta noi continuiamo a lavorare al Senato assiduamente, con grandi sacrifici, per poi non sortire alcun risultato, perchè è inutile passare ore e ore a parlare di questo provvedimento

denaro e di organizzazione, e naturalmente non potranno cambiare. Infatti, se anche emaniamo una legge più completa ma di fatto non coinvolgiamo nell'attuazione le Regioni, e man mano le istituzioni ai più bassi livelli, è tutto inutile perché sarà ancora peggio, soprattutto, quando presentate un testo unico largamente condivisibile ma senza una copertura fonanziaria sufficiente per poterlo attuare. Ragionate su questo. Parliamo di lavoratori atipici, parliamo di lavoratori interinali una volta per sempre perché sono una realtà. Se mi permettete,

grande esperienza e potrebbero contribuire tantissimo nel portare avanti queste idee. Non credo siano soltanto i sindacati o altri che sicuramente che sicuramente hanno grandi meriti, ma vi sono altre figure che si sono consolidate in questi anni, che fanno parte di un patrimonio che non si può disperdere. Per esempio, il medico competente che voi richiamate, come ha già detto la Commissione sanità: credetemi, quel quel parere non è stato stilato dal centro-destra o dall'opposizione, ma 13 punti a sfavore, 13 critiche ben precise - è chiaro che è stato stilato da una maggioranza, ma non è stato votato, come ripeto - mettono in evidenza, per esempio, la posizione proprio del medico competente; una figura che purtroppo non ha la stessa valenza istituzionale e professionale di altre professioni. Ecco perché vi chiedo un minimo di riflessione:

ha ragione la senatrice Pellegatta, che prima parlava, in termini molto impegnativi, della traccia di sangue che il nostro Paese porta nella sua storia del lavoro, però, è anche giusto collocare nel modo più corretto il vero significato di questa traccia dolorosa e la sua contestualizzazione ci aiuta a comprenderne davvero i confini e la portata. Va dunque ricordato che nel dopoguerra, cioè nella prima metà degli anni Cinquanta, si registravano ogni anno oltre 3.000 morti per infortuni sul lavoro.Questo dato si è poi trascinato fino agli Settanta, mentre dal 1975 il fenomeno ha cominciato lentamente, ma progressivamente a decrescere. Non è è difficile cogliere quanto su questo fronte abbia influito, dagli inizi degli anni Settanta, l'introduzione dello Statuto dei lavoratori.

e ad infortuni indennizzati, mentre i casi mortali, quelli che colpiscono di più e spesso fanno rabbrividire, sono 2,8 ogni 100.000 occupati in Italia, contro i 2,9 della media nell'Eurozona. L'Europa ci ricorda che creare un numero maggiore di posti di lavoro di migliore qualità è proprio l'obiettivo che l'Unione Europea si è data durante il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, quel Consiglio europeo che ha aperto la strada a una nuova visione delle politiche del lavoro, spostando l'accento dalle politiche passive a quelle attive e indicandoci non solo cifre da raggiungere, come per la maggiore occupazione (non solo con riferimento al tasso di occupazione, ma anche al tasso di occupabilità, concetto fondamentale che Lisbona introduce), ma anche l'elemento fondamentale chiamato qualità del lavoro, *more* *job* *and* *better* *job*, che è il secondo pilastro della Strategia di Lisbona. Certo, la salute e la sicurezza sono elementi essenziali della qualità del lavoro e rientrano tra gli indicatori adottati di recente anche dall'ultima comunicazione della Commissione europea, intitolata "Investire nella qualità". Noi, quindi, nel nostro Paese, all'interno dell'Unione Europea, possiamo presentare il bilancio positivo - lo ha ricordato bene prima di me il senatore Massidda - che la legge Biagi ha fatto emergere: una nuova conformazione del mercato del lavoro e la necessità di adeguare a tale nuova conformazione anche le forme di sicurezza,

In ogni caso, le cifre che oggi registriamo, soprattutto sul versante europeo, restano comunque alte, soprattutto in riferimento all'ingresso di nuovi Paesi, che su questo fronte ci portano - ahimè - un carico pesante da sopportare. I dati ci incoraggiano però anche a sviluppare una strategia più globale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, in quanto la qualità dell'occupazione consta di varie componenti solidali: solidali: tipo di qualifiche richieste per il posto di lavoro; livello di formazione dei lavoratori; natura del loro rapporto di lavoro; organizzazione del loro lavoro e dell'orario di lavoro. Se non si affrontano direttamente questi temi, è difficile svolgere e declinare quella promozione della salute sul luogo di lavoro che deve essere affrontata nel quadro dell'evoluzione generale delle attività economiche (più servizi rispetto al passato), delle forme di occupazione (maggiormente diversificate della popolazione attiva (che oggi è cambiata, con un maggior numero di donne che partecipano al mercato del lavoro, ma anche di lavoratori anziani) e della società in generale, maggiormente diversificata, ma sempre più contraddistinta da quell'esclusione sociale che tutti noi combattiamo e che l'Europa ci chiede di combattere. Un'organizzazione e un ambiente di lavoro sani e sicuri sono peraltro fattori che migliorano le prestazioni dell'economia e delle imprese. In effetti, le relazioni tra la salute sul luogo di lavoro e la competitività sono più complesse della semplice questione dei costi legati al rispetto delle norme. La "non qualità" del lavoro si traduce in una perdita di capacità produttiva per l'economia e in spese per indennizzi e prestazioni, il cui finanziamento pesa, in larga misura, sulle imprese. Al di là, quindi, dei drammi di natura umana, si tratta di uno spreco di risorse nel contesto dell'invecchiamento strutturale della popolazione attiva. A livello dell'impresa stessa, la "non qualità" si traduce in un degrado della sua immagine nei confronti del mondo esterno: dei dipendenti, dei clienti, dei consumatori e più in generale del pubblico, sempre più sensibile ai temi legati alla sicurezza. Ecco perché, secondo noi, su questo crinale della sicurezza sul luogo di lavoro si gioca una delle sfide della responsabilità sociale delle imprese nei confronti dei propri *stakeholders*. Un ambiente di lavoro sano consente, inoltre, di affermare l'immagine di prodotti o di servizi di qualità e il suo miglioramento dipende da una strategia globale di "gestione della qualità" e di responsabilità sociale che apporta benefici alle prestazioni, in modo particolare alla competitività. L'economia della conoscenza, che Lisbona considera il cuore di una nuova strategia economica e sociale, è contrassegnata da trasformazioni profonde che riguardano la società, l'occupazione e gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Noi pensiamo, ad esempio, che il lavoro svolto nella passata legislatura ad iniziativa del Governo Berlusconi sia ancora molto valido. Le ragioni delle scelte elaborate con il testo proposto nella passata legislatura mantengono tutta la loro piena validità, in primo luogo in relazione all'esigenza di pervenire finalmente al coordinamento e alla semplificazione di un sistema normativo che si è sedimentato nell'arco di un cinquantennio e del quale si rende necessario assicurare l'operatività, a fronte di quella ineffettività che si è riscontrata soprattutto negli ultimi anni. Tale ineffettività è il problema principale da combattere e il legislatore è chiamato ad affrontare i motivi per cui si sono resi inefficaci ed ineffettive queste leggi. La disciplina vigente in materia di sicurezza del lavoro è stata infatti elaborata, secondo noi, con riferimento alle imprese di grandi dimensioni e si fonda pertanto su un approccio prescrittivo supportato da adempimenti di carattere formale, con un elevato livello di burocratizzazione. Questa impostazione si è rivelata del tutto inefficace nei confronti delle piccole e medie imprese e, più in generale, di una realtà del sistema produttivo italiano caratterizzato da un forte decentramento, quando non di un vero e proprio policentrismo legato all'economia dei distretti. Occorre quindi, secondo noi, mutare la filosofia stessa del sistema normativo in materia di sicurezza sul lavoro e dare vita ad un testo unico la cui effettività nei confronti della piccola impresa sia garanzia di effettività anche nei confronti dell'impresa di grandi dimensioni e che si deve connotare, in primo luogo, per certezza e semplicità della norma, come presupposto vitale per la sua applicabilità. A tal fine, secondo noi, è essenziale l'adozione di un approccio sostanzialistico e per obiettivi, oltre le forme e i formalismi, con alcune caratteristiche specifiche. In primo luogo, occorre prevedere che le funzioni pubbliche nel campo della sicurezza sul lavoro possano essere svolte con il concorso delle parti sociali, in un rapporto fondato sul principio di sussidiarietà, anche traendo spunto dalle positive esperienze di bilateralità realizzate con grande successo nel settore dell'edilizia e dell'artigianato. D'altra parte, è innegabile che un vero ed effettivo incentivo alla bilateralità presuppone che, laddove essa si afferma, si realizzi una proporzionale riduzione degli adempimenti e dei controlli. Un altro problema al quale secondo noi è urgente trovare una positiva risoluzione nel testo unico riguarda l'esigenza di individuare modalità operative condivise con le Regioni per superare le ambiguità della disciplina costituzionale che, come è noto, ha alimentato a dismisura il contenzioso innanzi la Corte costituzionale. A noi, quindi, pare di poter dire, con grande forza, che il nostro giudizio negativo su questa proposta è legato fondamentalmente alla somma dei tanti fattori normativi che aumenteranno a dismisura burocrazie e rigidità a perdere di vista la sostanziale efficacia di una normativa che dovrebbe guardare di più e meglio nel particolare e nel sistema economico italiano così frammentato salvaguardare un principio, ossia che ciò che conta è il risultato che noi vogliamo ottenere. E non lo otterremo in virtù di un approccio solo formale e ideologico, attraverso balzi, balzelli e nuove burocratizzazioni, ma - anzi - faremo sì che quel lavoratore sarà sempre meno protetto, invece che più protetto, nella sostanza dei fatti, al di là delle parole, signor

Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni politiche su questo provvedimento e su come esso è arrivato alla nostra attenzione e all'attenzione della pubblica opinione.

e, come sempre accade in questi casi, ne è nato un moto di opinione mediatica che ha portato innanzitutto i principali sindacati a dedicare la giornata del 1° maggio di quest'anno proprio a tale tema

oppure si fa una legge, che resta come una grida manzoniana. In questo modo, nominando una Commissione o facendo quella legge, si tacita l'opinione pubblica che è stata sollecitata a ritenere che il problema fosse di grave emergenza e fosse quindi stato affrontato. Ebbene, in questo caso abbiamo fatto l'una e l'altra cosa: abbiamo istituito una Commissione d'inchiesta che analizzasse il problema e stiamo facendo una legge per rispondere all'emergenza, ma se guardiamo i dati forse ci rendiamo conto che il problema esiste ma non è di così grave emergenza. Premetto, signor Presidente, a queste mie considerazioni il fatto che sono tra i presentatori, assieme ai colleghi Sacconi, Gentili, Morra, Novi e Piccone, sui luoghi di lavoro e quindi non rappresento qui la voce di quelli insensibili ad un tema grave o che considerano gli incidenti sul lavoro una grave fatalità a cui rassegnarsi. Sono, al contrario, dell'opinione che bisogna arrivare, come ha detto oggi in Aula il collega Zuccherini, ad un modello organizzativo del lavoro

si sono mantenuti stabili gli incidenti sul lavoro e gli incidenti mortali, si potrebbe pensare che non abbiamo fatto un passo avanti. Ciò varrebbe se si fossero mantenuti stabili in termini assoluti,

a fronte di un mercato del lavoro che dà impiego ad un numero maggiore di persone, corrisponde in realtà ad una tendenza progressiva al calo degli incidenti sul lavoro. Se poi andiamo ancora più nei dettagli, ci accorgiamo che, su 1.376 incidenti mortali circa 850 sono frutto di una sola causa: si collocano nel settore dell'edilizia e sono determinati dalla caduta dalle impalcature (su questo vorrei svolgere poi qualche considerazione) e che un'altra parte consistente di essi in realtà non sono incidenti veri e propri nello svolgimento della mansione lavorativa da parte di chi sta facendo un lavoro, ma avvengono negli spostamenti da un luogo di lavoro all'altro, da uno stabilimento all'altro, da un cantiere all'altro e questi, seppur rubricabili come incidenti che si svolgono durante l'orario di lavoro e nello svolgimento di mansioni lavorative, non sono attribuibili alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature di lavoro, ma al problema della sicurezza delle nostre strade e quindi andrebbero affrontati non con una normativa specifica sugli incidenti sul lavoro ma, in termini più generali, rinnovando le nostre infrastrutture, le nostre strade e potendo contare su strade che offrano una sicurezza di natura passiva, passiva, come si dice, maggiore rispetto a quella attuale. Se allora derubrichiamo questa parte di incidenti sul lavoro e consideriamo la grande rilevanza degli incidenti in edilizia che nascono dalle cadute dalle impalcature,

costante ricorrenza di un atteggiamento pericoloso della società italiana, ossia quello di sollevare allarmi ed emergenze, adottare leggi di carattere emergenziale e poi infischiarsene - mi scusi, Presidente, per il termine poco

nessuno di tali lavoratori è morto perché mancava la norma che imponeva un determinato atteggiamento di sicurezza, una strumentazione adeguata o una preparazione professionale di un certo tipo. accade perché i controlli non sono penetranti o non lo sono sufficientemente. Di chi è, signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, la responsabilità del controllo amministrativo se non del Governo?

«geolegislatori»: ormai siamo al carotaggio nell'archivio di Stato, per capire il numero e gli strati di leggi che si sono addensati sulla Repubblica italiana. Aggiungeremo una nuova delega legislativa e nuovi decreti delegati, che non porteranno un'oncia di beneficio e alcun miglioramento nella situazione; al contrario, si aggraverà la situazione di molte imprese e di molti lavoratori e probabilmente vi sarà un ulteriore effetto dissuasivo sulla creazione di posti di lavoro e un sicurissimo effetto dissuasivo sull'emergere del lavoro sommerso. sommerso. Signor Presidente, dobbiamo dircelo con chiarezza: la maggior parte degli incidenti in edilizia avvengono non nelle imprese che operano nel pieno della trasparenza e della legalità e che rispettano la legislazione, bensì nelle imprese che sono in qualche modo sommerse, che usano il lavoro nero e che sono fuori dal perimetro della legalità.

e invece lavorano. Il problema sarebbe tutto del Governo e della sua capacità di far funzionare l'apparato amministrativo. Siccome il Governo è in tutt'altre faccende affaccendato, della funzionalità dell'apparato amministrativo poco si occupa e ci offre dunque questa grida manzoniana di cui poco abbiamo bisogno. Detto questo, Presidente, vogliamo anche adottare un cambiamento di mentalità nell'approcciare questi temi? Sono circa trent'anni che sto

alle quali le imprese sono, di per sé, entità del male, non hanno nessuno rispetto della vita delle persone e, in questo caso, della sicurezza delle persone e non hanno alcuna considerazione perché, se muore un lavoratore, tanto lo si può sostituire. Così si rappresenta spesso il mondo delle imprese. Non è per nulla vero. Io non conosco un'impresa dove sia considerato irrilevante anche il pur minimo incidente sul lavoro, intanto perché dal punto di vista umano è un problema per chiunque ed io non conosco imprenditori che non abbiano alcuna sensibilità per i loro collaboratori, ma in secondo luogo perché, anche volendo tacciare di massimo cinismo l'imprenditore dedito solo a a contabilizzare il suo profitto - situazione che esiste solo in una certa fumettistica di sinistra - la verità è che si produce un danno economico per l'impresa se un lavoratore capace, esperto, competente, che sa far funzionare l'apparecchiatura cui è destinato, che sa far andare avanti la produzione si ferisce in maniera anche grave e deve abbandonare, magari per un lungo periodo il posto di lavoro. Inoltre, è un danno economico per la collettività, se questo incidente si riflette poi su costi complessivi nel prestare cure, riabilitazioni e altri servizi assolutamente indispensabili che vanno prestati. È quindi interesse comune dell'impresa come dei lavoratori che gli incidenti siano minimizzati, perché essi gravano sui bilanci delle imprese e sui redditi di tutti come un costo aggiuntivo e non come un incidente irrilevante o una variabile indipendente della produzione (tanto per parafrasare un linguaggio che un tempo attribuiva al salario questa caratteristica, in quanto variabile indipendente rispetto alla produzione di ricchezza).

Ci sono numerosissimi casi di infortuni sul lavoro, in particolare nel campo dell'edilizia - signor Presidente, signor rappresentante del Governo - dove la responsabilità è tutta - ahimé - spesso in capo a chi l'incidente, poi, lo subisce. Io ho conoscenza diretta di questo settore, perché un mio stretto parente è architetto, è responsabile della sicurezza del lavoro nei cantieri, ha dovuto seguire un corso di abilitazione per conseguire questa qualifica ogni volta che si apre un cantiere per una costruzione o una ristrutturazione lui predispone tutta la strumentazione necessaria per garantire la sicurezza ai lavoratori (elmetti, imbragature, ganci di sicurezza, scarpe rinforzate e così via), e svolge a tutti i lavoratori un breve corso sull'utilizzo di queste dotazioni, controllando che siano utilizzate. Ma dirò di più. Quando lui va in cantiere (vestito un po' come noi, in giacca e cravatta), indossa le scarpe rinforzate di acciaio, l'elmetto e se sale su un'impalcatura si imbraga e si lega con i moschettoni

che nel *box* di casa sua ha esposto, come in una bellissima galleria, gli elmetti di tutti i cantieri significativi che ha gestito nella sua attività professionale, ognuno con un colore ed una scritta diversi legati all'impresa presso cui in quel momento svolgeva il lavoro.

tutte le dotazioni vengono immediatamente dismesse dagli stessi lavoratori a cui lui ha minacciato sanzioni disciplinari anche gravi nel caso in cui le avessero dismesse: i lavoratori, insomma, si tolgono l'elmetto perché fa caldo e dà fastidio, si staccano l'imbragatura perché fa lavorare più lentamente, si sfilano le scarpe di sicurezza perché sono pesanti e fanno male e, grazie a Dio, nel 99 per cento dei casi, non accade nulla, se non magari qualche chiodo che si infilza sotto la pianta del piede per mancanza di attenzione. attenzione. Ma noi consideriamo tutto questo nel provvedimento al nostro esame? No. Il lavoratore è trattato come un bambino irresponsabile a cui al massimo dobbiamo fare corsi.

spaventose, minacce di licenziamento o altro, ma basterebbe sapere che, se arriva l'ispettore del lavoro, c'è la multa all'impresa ma anche la multa di 50 euro a ciascun lavoratore

non consideriamo le situazioni reali, calcoliamo gli incidenti stradali come fossero incidenti sul lavoro laddove i problemi sono le infrastrutture alla viabilità e facciamo una bella grida manzoniana senza controllare.

e le aziende in veri e propri cantieri pieni di cartelli, di indicazioni, di piste, manca solo il *briefing* iniziale come sugli aerei, quando parte il filmato e l'assistente di volo illustra come indossare il giubbetto di salvataggio o indica il corridoio luminoso verso le uscite di sicurezza. Ci rendiamo ridicoli di fronte al Paese e graviamo le imprese

*c)*, si legge: «applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (...) prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; (...)». In poche righe

*e**)* del comma 2 dell'articolo 1, che recita: «riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo». Anche in questo caso si tratta di una materia vastissima, che credo verrà affrontata con centinaia di articoli, anche perché spero che non si torni,

che le leggi siano fatte bene, ma al termine del mio intervento tornerò su un punto che dimostrerà che delegare al Governo, privando di fatto il Parlamento di quella facoltà e di quel dovere di fare le leggi e di controllare, ma in modo reale, gli atti del Governo (figuriamoci quando il Governo agisce in via del tutto straordinaria, dice la Costituzione, per redigere lui stesso le leggi), non sempre è positivo. Intanto rivolgo un invito al rappresentante del Governo e, attraverso lui, in particolare al Ministero

dunque un esplicito invito al Governo a risponderci su questo punto. Intervengo poi su due aspetti specifici di questo provvedimento. Il

lavoro. Forse che una strumentazione o un ambiente di lavoro che può essere salubre per un italiano può non esserlo per un immigrato o viceversa? Forse che se un immigrato cade non si fa male esattamente come un italiano?

«Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192,» (un comma che incoraggia - e questo va benissimo - la regolarizzazione

anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori». Qui si sono criticate le sanatorie, i condoni del Governo Berlusconi,

che per un anno non si facciano i controlli sulla tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. È una cosa spaventosa! Ecco perché non bisogna abdicare alla nostra facoltà

sul quale esprimo tutte le mie perplessità riallacciandomi all'intervento di diversi colleghi? Facciamola questa cosa e ricordiamoci che, se ci fosse stato un aumento degli infortuni (che, mi pare, grazie al cielo non c'è stato, probabilmente perché nessuno

pagare per regolarizzarli (e questa è una buona cosa), ma per un anno, pazienza, non si sarebbero fatti più i controlli sulla sicurezza. È veramente una cosa incredibile che ci consiglia una volta di più di non fidarci del Governo per fare le leggi, anche perché è nostro dovere, ce lo dice la Costituzione che dobbiamo farle noi le leggi e non lasciare che si facciano queste mostruosità che, ripeto, nessun senatore, né dell'opposizione, che ha votato contro, ma neanche della maggioranza, costretta a votare a favore per via del voto di fiducia - cosa che non li esenta dalle loro responsabilità ma diciamo che li giustifica - avrebbe mai accettato. *(Applausi dal Gruppo

Presidente, mi consentirà di iniziare con una breve battuta polemica nei confronti del senatore Stracquadanio. Credo sia molto arduo tentare di dimostrare che che gli incidenti sul lavoro abbiano una rilevanza inferiore rispetto ai dati che tutti conosciamo perché molti incidenti avvengono durante il percorso tra la casa e il lavoro o da un posto di lavoro all'altro. È esattamente il contrario, e questo lo dimostra spesso la magistratura, ma per non ricorrere alla magistratura basta leggere i risultati delle indagini svolte in questi anni.

che l'incidenza degli infortuni sul lavoro è più bassa utilizziamo altri dati, non raccontiamo queste storielle perché non riguardano assolutamente la storia di questo Paese. Vi è una conclusione comune riguardo all'esigenza di un intervento organico su queste materie che deriva dalle varie Commissioni d'inchiesta che si sono succedute in questi ultimi 15-20 anni. Ho avuto modo di leggere la relazione conclusiva della Commissione Lama, poi della Commissione Smuraglia, poi della stessa Commissione Tofani

Ed è evidente, senatore Malan, che se occorre un intervento di riordino e di razionalizzazione, bisogna procedere attraverso una delega. Questo lo avete fatto anche voi nella passata legislatura: il Governo il Governo chiedeva una delega al Parlamento per poter intervenire su questa materia. Quando ci sono interventi di questa complessità si opera in questa direzione, si fa così: non c'è un altro modo.

presenta delle sue valutazioni e il Parlamento deve intervenire sui criteri direttivi - come succede sempre perché il controllo parlamentare si deve esercitare in questo modo - il Governo non è stato fermo in questi mesi e in questo anno

Si è introdotta una norma per garantire più sicurezza nelle gare di appalto. Quindi, è vero che si produce una delega; è vero che la delega avrà i suoi tempi d'attuazione per l'emanazione dei decreti legislativi, ma nello stesso tempo il Governo è intervenuto - credo - giustamente attorno alle questioni più rilevanti dal punto di vista dell'emergenza. È anche vero - e questo mi dispiace dirlo, ma l'ho già ricordato anche in altre occasioni - che alcune previsioni della legge finanziaria (per esempio il taglio orizzontale su tutti i Ministeri) a volte producono dei danni. Penso agli ispettori che non hanno i mezzi e le attrezzature per poter uscire e condurre le ispezioni perché appunto si sono ridotti gli stanziamenti a loro destinati. C'è un dato - voglio ricordarlo - emerso anche nella relazione conclusiva della Commissione presieduta dal senatore Tofani nella passata legislatura: passata legislatura: moltissimi degli incidenti del lavoro si verificano in capo ai cosiddetti lavoratori precari; questo genere di lavoratori perché c'è poca informazione, poca prevenzione e poca formazione, appunto perché trattandosi di rapporti di lavoro precari non si investe per garantire la sicurezza. È la solita logica competitiva che abbassa i costi del lavoro, ma è anche la logica che crea una concorrenza sleale nel mercato del lavoro tra le aziende che rispettano tutte le norme e quelle, invece, che non le rispettano. Allora, Allora, ritengo - non lo dico in termini polemici - che sarebbe necessario un confronto vero. Il presidente di Confindustria dice che questa situazione è intollerabile, che vuole avere un rapporto con il mondo del lavoro e con le organizzazioni sindacali per trovare insieme le soluzioni. La prima strada che bisogna imboccare è proprio questa: cercare di evitare che le storture previste dalla cosiddetta legge n. 30 del 2003, la legge che ha aumentato le flessibilità e precarietà nel mondo del lavoro, possano produrre l'aumento degli incidenti sul lavoro. Questa è una questione che

presieduta dal presidente Tofani, un senatore di Alleanza Nazionale, che dice esattamente questa cosa. Dice che la stragrande maggioranza degli incidenti avviene in quei posti dove ci sono rapporti di lavoro precario. precario. Credo che questo sia un tema da affrontare. Occorre ovviamente più informazione, più formazione, più prevenzione, più repressione; occorrono norme più snelle, che facilitino la loro applicazione e la loro efficacia.

importante nell'obbligo della presentazione del documento sui rischi che deve essere discusso, trasparente e conosciuto da parte di tutti i lavoratori. Un ruolo altrettanto importante è rivestito dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che devono essere più autonomi, devono avere più poteri, più autonomia nella possibilità di intervenire sui processi produttivi facendo proposte. Occorrono norme più precise, più trasparenti per garantire la loro elezione, che deve venire dai lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza non devono essere indicati dalle organizzazioni sindacali; devono essere eletti dai lavoratori. Ovviamente, come dicevo prima, stiamo discutendo di una delega al Governo che quindi avrà i tempi necessari per poter essere

dalla Commissione Smuraglia alla Commissione Tofani - è che occorre più coordinamento tra le varie attività ispettive. È di certo una questione delicata perché devono convivere le competenze delle Regioni

al rispetto e alla tutela dell'ambiente. La materia è molto complessa e però uno dei dati fondamentali è riuscire a garantire più coordinamento e più efficacia nelle varie attività ispettive.

e già da tempo finalizza una quota del proprio bilancio alla incentivazione di misure per garantire la sicurezza nei posti di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese. Occorrono forme di incentivi per stimolare le aziende a praticare le migliori disposizioni e pratiche scientifiche più avanzate. Bisogna Bisogna stimolare le aziende, per esempio valorizzando gli accordi aziendali che prevedono misure per migliorare la sicurezza e, a mio avviso, in questo campo serve anche il cosiddetto valore dell'esempio virtuoso. signor Presidente, ritengo che abbiamo corso negli anni passati un rischio importante perché le norme sulla sicurezza devono essere unitarie e valere su tutto il territorio nazionale. Devono valere in Sicilia

quando si è trattato di riformare il Titolo V della Costituzione, quando si prevedeva di inserire questa materia della sicurezza tra quelle concorrenti tra lo Stato e le Regioni. Avevamo commesso un errore, che è stato superato perché - ripeto -queste norme devono valere in modo unitario su tutto il territorio nazionale. la delega che stiamo esaminando, augurandoci che venga approvata nel più breve tempo possibile dai due rami del Parlamento. *(Applausi Presidente, colleghi, innanzitutto consentitemi di richiamare alcuni dati, soprattutto quelli relativi al *trend* di medio periodo, che si può evincere confrontando il periodo 2002-2006 secondo quanto ci dice l'INAIL. In questo arco temporale si registra una riduzione complessiva del numero di infortuni del 6,5 per cento nel corso di questo quinquennio, cioè dai 993.000 infortuni del 2002 ai 928.000 del 2006. E ancora più sostenuto è il calo degli infortuni mortali che, considerando per il 2006 una stimadel dato consolidato, si attesta comunque attorno al 10 vale a dire un risparmio annuo di circa 150 vite umane nel 2006 rispetto al 2002. In termini relativi, rapportando cioè gli infortuni alla forza-lavoro che li esprime e tenendo conto che l'occupazione è cresciuta del 4,9 per cento nel quinquennio, la contrazione infortunistica, espressa dai tassi di incidenza, risulta più sostenuta e significativa sia per quanto riguarda gli infortuni nel loro complesso (- 10, che per i casi mortali per i quali il dato 2006 consolidato si stima comporterà una riduzione nell'arco del quinquennio nell'ordine del 15 Il secondo dato che voglio considerare è quello comparato con gli altri Paesi europei. Il nostro Paese presenta per gli infortuni nel loro complesso un indice pari a 3.085 infortuni per 100.000 occupati, al di sotto sia del valore riscontrato per l'Eurozona (3.698) sia per quello dell'Unione Europea dei quindici (3.221). La graduatoria risultante dalle statistiche armonizzate colloca, quindi, l'Italia anche per il 2004 ben al di sotto di Paesi assimilabili al nostro come Spagna, Francia e Germania. Per i casi mortali l'Italia, con un indice nazionale di 2,5 decessi per 100.000 occupati, si colloca perfettamente in linea con il dato rilevato per i 15 Stati membri e al di sotto di quello registrato nell'Eurozona del 2,8, che comprende Paesi più omogenei al nostro sia dal punto di vista dei sistemi assicurativi sia di quello della omogeneità e completezza dei dati. Ho sostanzialmente citato, come ho detto, la fonte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. è giusto riportare il problema alle sue esatte dimensioni ma, allo stesso tempo, mantenere doverosamente alta l'attenzione morale prima ancora che politica per contrastare un fenomeno che, se solo anche producesse una vittima, dovrebbe indurci a rafforzare i presidi che possono prevenire il formarsi del danno per una persona al lavoro. Hoalcuni ricordi della trascorsa legislatura. Iniziammo la legislatura, affidando al professor Marco Biagi un Libro bianco sul mercato del lavoro ed egli, in quell'ambito, dedicò alla patologia degli infortuni sul lavoro una specifica attenzione, individuando sostanzialmente tre problematiche. un eccesso di regolamentazione quale si è prodotto per il recepimento di numerose direttive via via accumulatesi e sedimentatesi sopra il fondamentale decreto legislativo n. 626 e tutta la produzione normativa precedente degli anni Cinquanta, Cinquanta, con il risultato quindi di un'incertezza della norma e di una sua diffusa ineffettività. In secondo luogo, una mancanza di buone prassi e di criteri prevenzionistici specifici per le piccole imprese e per l'agricoltura, perché, nel complesso il nostro assetto regolatorio è tutto orientato sulla media, medio-grande e grande impresa strutturata e trascura quella grande dimensione del nostro sistema produttivo, nella quale peraltro si concentra larga parte degli infortuni, composta da imprese diffuse, spesso sommerse, che operano in particolare nell'agricoltura, nell'edilizia e nei servizi. Il terzo problema che Marco Biagi segnalò era quello dei nuovi lavori, dei cosiddetti lavori atipici (che in realtà sono sempre più tipici di un mercato del lavoro che cambia), e del lavoro autonomo, che nel nostro ordinamento ancora oggi è sottratto a ogni disciplina relativa alla salute e alla sicurezza nel lavoro. Non è un caso che proponemmo subito all'esame del Consiglio dei ministri e poi del Parlamento un complesso di norme delega inserite nel disegno di legge di semplificazione, che furono approvate nel 2003 con il voto contrario dell'opposizione, un voto accompagnato da aspre polemiche, che segnarono un radicale conflitto tra maggioranza e opposizione, anche se accompagnato dal consenso di tutte le organizzazioni dei datori di lavoro, dal commercio all'artigianato, all'agricoltura, all'industria, da un atteggiamento dialogante di CISL e UIL e, come al solito, dal conflitto radicale con la CGIL, sulla quale normalmente si tarava, come si tara ancora oggi, la coalizione di centro-sinistra. Producemmo il decreto delegato che ora è oggetto del disegno di legge a firma mia e di altri colleghi, il cui esame è abbinato a quello del disegno di legge del Governo

una rigida interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione, che noi cercammo inutilmente di cambiare, laddove lo stesso prevede, con una definizione assolutamente incerta nella sua interpretazione, la tutela e la sicurezza del lavoro materia di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Ci fu allora un parere del Consiglio di Stato, che segnalò alcuni criteri

che a noi chiesero rigidamente, un interpretazione a mio avviso pericolosa, quella secondo la quale avremmo dovuto dar vita a tanti sistemi della sicurezza per ciascuna Regione, rendendo ancor più difficile l'obiettivo della effettività delle norme, già oggi reso complesso dalla loro incerta interpretazione. Peraltro, non ci limitammo a questo. Nella trascorsa legislatura producemmo un atto importante, la legge Biagi, quella che vi ostinate a chiamare con un numero, perché probabilmente avete bisogno di sciacquarvi la bocca prima di nominare il nome di Marco Biagi. La legge Biagi si preoccupò di estendere a tutti i lavori le tutele, cosa che poi ritornava nel nostro provvedimento, nel decreto delegato, che però considerava doversi applicare le nuove disposizioni a tutti coloro che a qualunque titolo si trovano in un ambito lavorativo. La legge Biagi già prevedeva però tutele fondamentali e quindi incrementava il grado di protezione dei nuovi lavori, nella convinzione che si dovesse così anche preparare l'auspicato, da Marco Biagi come da noi, Statuto dei lavori, fondato su una base di tutele sostanziali L'altra novità che introducemmo fu quella relativa alla riforma dei servizi ispettivi centrali, cioè l'integrazione dei servizi ispettivi dell'INPS, dell'INAIL e del Ministero del lavoro - compreso il Nucleo dei Carabinieri che operano, da allora, doverosamente in modo integrato, cioè, comunicano l'uno all'altro le attività ispettive ed operano insieme, ciascuno per le proprie competenze, dando così ai circa 6.000 ispettori una capacità operativa straordinariamente superiore rispetto al tempo nel quale essi operavano in modo assolutamente disgiunto l'uno servizio dall'altro. Aggiungo che demmo luogo al concorso per oltre 800 ispettori, solo in parte assunti, e qui si discute dei modi con i quali garantire la totale assunzione dei 600 circa che ancora, pur pur idonei, non sono stati assunti. Tuttavia, il tema del testo unico rimaneva necessariamente aperto. Bloccati noi dal conflitto con le Regioni, è stata cosa buona e giusta l'aver riproposto una legge delega per il testo unico e noi abbiamo condiviso questa necessità. Non occorreva una specifica enfasi su un fenomeno che è sempre stato, fortunatamente, all'attenzione del Governo e del Parlamento per affermare l'esigenza di un testo unico che desse maggiore effettività alle norme attraverso una maggiore certezza. Voglio ricordare che noi abbiamo voluto sostenere questa maggiore certezza con un emendamento recepito dalla Commissione nel corso suoi lavori, quello in base al quale si estende anche alle norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro il cosiddetto diritto d'interpello che noi abbiamo già introdotto con la legge Biagi, quello per il quale alcuni soggetti a ciò abilitati (come le associazioni di rappresentanza) possono chiedere ed ottenere con certezza e in tempi brevi una interpretazione autentica da parte del Ministero del lavoro (in questo caso di una Commissione, che mi auguro sarà definita in modo semplice, comprendente Regioni, Ministero del lavoro e Ministero della salute). La risposta all'interpello consente, infatti, certezza a tutti gli interpreti e a a coloro che sono preposti ad applicare la norma, ma anche ai servizi ispettivi che devono evitare un florilegio interpretativo che crea disordine e non aiuta l'obiettivo di produrre sicurezza. Tuttavia, il vostro disegno di legge ha un difetto fondamentale: si muove, cioè, sulla base di un presupposto opposto a quello che noi avevamo adottato. Noi partivamo dall'idea che era di Marco Biagi, il quale, tra tra le moltissime cose che ha depositato, aveva lasciato anche un robusto lavoro per la produzione di questo testo unico. Marco Biagi era solito dire (e lo diceva in inglese, amando la sostanzialità del *common law*): law*): *management by objectives but not by regulation*. Chiedeva, cioè un approccio per obiettivi e non per regole, o più per obiettivi che per regole, cioè un approccio non formalistico, ma sostanzialista, un approccio che consentisse di contrastare le patologie nei luoghi di lavoro e tutto ciò che mette a repentaglio l'incolumità della persona al lavoro attraverso strumenti strumenti che consentissero di raggiungere risultati. L'ansia di Marco Biagi, in generale, era l'ansia del riformista che vuole risultati, che non accontenta la propria coscienza attraverso il deposito di una norma, magari astrusa, che si rivela ineffettiva nella realtà. Egli era fortemente dall'ansia di vedere gli effetti risultati dalle norme alle quali lavorava. E questo approccio caratterizzò la nostra proposta quanto voi rimanete, più che mai esasperate la vecchia impostazione che vuole contrastare il fenomeno degli infortuni nel lavoro attraverso adempimenti formali esasperati sostenuti da sanzioni ancora più enfatizzate, con il risultato che proprio nella dimensione nella quale gli infortuni più si producono questo combinato disposto non genererà effetti, non ne produrrà. Pensate alla alla sospensione dell'attività di impresa. Quando quell'impresa è precaria, è sommersa o emersa solo per una parte, non si preoccupa della sospensione dell'attività, muore e rinasce sotto altre forme, con la flessibilità che è tipica dell'attività sommersa, ma potreste mettere a repentaglio terzi incolpevoli, come i lavoratori, attraverso la sospensione dell'attività d'impresa anche solo per eccesso di ricorso alle ore straordinarie, che si produce tipicamente nelle realtà nelle quali vi è carenza di manodopera, in cui le parti, colludendo (non giustamente: non voglio con ciò giustificarle), talora pur di completare un'opera magari ricorrono esageratamente al lavoro straordinario. Quella sanzione sarebbe la sospensione dell'attività d'impresa, che in generale abbiamo contestato ovunque sia stata proposta, proprio perché colpisce i terzi incolpevoli. Oppure, penso alla responsabilità oggettiva che caricate sugli amministratori, fino ad al punto della loro interdizione dalle funzioni amministrative, di fronte a reati che sarebbero colposi e non dolosi come sono quelli per i quali questa responsabilità è stata sin qui introdotta. O ancora, quando pensate di separare l'arresto dall'ammenda, con ciò facendo venire meno quell'obiettivo, sempre sostanziale, di stimolare il ravvedimento operoso, che è sostenuto ovviamente dal pagamento dell'ammenda in luogo dell'arresto, ravvedimento che ci interessa molto di più che non la soddisfazione dell'arresto, perché ci interessa rimuovere le ragioni che possono generare il danno ad un lavoratore. L'apparato sanzionatorio, quindi, non è casuale: è conforme ad un approccio tutto esasperatamente formalistico, che oltretutto si tara ancora sempre sulla grande impresa, alla quale volete anche associare il lavoro autonomo non nelle forme circoscritte che avrebbero rappresentato un passo avanti rispetto alla disciplina precedente, ma allo stesso tempo verosimile e coerente con la natura del lavoro; noi che il lavoro autonomo dovesse essere richiamato all'uso dei dispositivi di protezione individuale e alla sorveglianza medica periodica, voi, con una delega molto ambigua a questo riguardo, lasciate intendere che il lavoro autonomo potrebbe entrare nel complesso delle disposizioni, come ho detto, ancor più "starate" rispetto alle sue caratteristiche perché disegnate sulla grande impresa strutturata, quel modello ideale al quale vi richiamate, come fa anche il ministro Visco, che ritiene la piccola, la microimpresa una patologia del nostro sistema produttivo che deve essere rimossa quanto prima e devo dire che qui dei contributi alla rimozione delle piccole imprese ci sono. Noi invece proponiamo un'altra strada: un approccio

in modo che, in quanto sistema di monitoraggio condiviso, consenta insieme di condividere la necessità di rafforzare i presidi in un settore, in un'area, in un ambito, piuttosto che in un altro, e quindi di correggere, aggiustare flessibilmente il tiro dell'azione positiva per raggiungere risultati e misurare quindi le politiche, le azioni, le stesse norme che devono sempre essere ritenute reversibili sulla base dei risultati che si conseguono. Cominciamo a governare, cioè, secondo una logica di quantistica che ci consenta di stabilire se l'azione è giusta o meno sulla base dei numeri, così come abbiamo cercato di fare con i tassi di occupazione ma, come ho detto prima, anche con i tassi relativi agli infortuni nel corso del passato quinquennio.

che venga ripreso quello strumento presso l'INAIL, consistente nel fondo a ciò dedicato. L'uso delle norme di buona tecnica e delle buone prassi deve essere sostenuto però dalla scelta del potere di disposizione da parte delle attività ispettive, soprattutto per le normative vecchie ed obsolete, che riguardano tecnologie Quanto è più importante cancellare tali norme e dare invece ai servizi ispettivi il potere di disposizione che chiede quando intervengono le tecnologie più moderne e la sanzione penale interviene solo dopo, quando quella disposizione non viene accettata ed adempiuta.

Proprio noi lo abbiamo sottolineato con forza pensando all'agricoltura, all'edilizia, all'artigianato, ambiti nei quali la bilateralità ha già, per fortuna, una grande funzione e ancora più grande ne può avere, ossia la produzione di organismi bilaterali, espressioni delle parti sociali. Là dove la bilateralità esiste e crea quindi il cono di luce di una forma di controllo sociale, perché non semplificare drasticamente, posto che le parti sociali insieme, concordemente, non possono che avere un approccio sostanzialista sostanzialista e molto migliore dell'approccio freddo e lontano dell'amministrazione, che chiede soltanto adempimenti formali? Alla bilateralità dobbiamo dare poteri e fare in modo che la sua attività ispettiva e di vigilanza possa dare luogo ad una certificazione.

che l'impresa deve essere l'epicentro del conflitto sociale e non il luogo della naturale e fisiologica cooperazione fra le parti, soprattutto quando è in gioco la salute del lavoratore e, più in generale, lo sviluppo della risorsa umana. Voi partite dall'idea che si deve invece incoraggiare il conflitto e tutto ciò che contrappone il lavoro e l'impresa; questo è un approccio che purtroppo non aiuta soprattutto i lavoratori.

il disegno di legge che stiamo discutendo è teso a definire un nuovo assetto complessivo della disciplina in un settore particolarmente delicato, quello della sicurezza sul lavoro, che ancora oggi, purtroppo, continua ad essere uno dei temi drammatici che la cronaca non smette di portare in evidenza quasi ogni giorno. Ogni anno mediamente il 6 per cento dei lavoratori italiani subisce un incidente sul lavoro. Si tratta di quasi un milione di incidenti di diversa natura e gravità, dei quali circa 600.000 con esiti di inabilità superiore a tre giorni; oltre 27.000 determinano una invalidità permanente nella vittima, e più di 1.300 ne causano la morte. Ciò equivale a dire che ogni giorno tre persone perdono la vita per disgrazie legate alla propria attività lavorativa. Il decreto legislativo n. 626 del 1994 è stato una tappa fondamentale per far crescere e maturare una coscienza critica circa tale problematica, introducendo innovazioni nel campo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, focalizzando l'attenzione sulle regole e gli strumenti operativi. Tuttavia, essa ha fallito nel suo obiettivo principale a causa della poca praticità di applicazione, degli eccessivi adempimenti formali, della frammentazione delle norme e delle disposizioni tecniche, della forte disorganicità. Già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva lavorato ad un Testo unico delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, poi arenatosi nel confronto con le Regioni, come ha ricordato il collega Sacconi. Ciò è comprensibile quando, dall'altra parte, si utilizzano le istituzioni per ostacolare un Governo avverso, pratica che non abbiamo mai compiuto e a cui mai ricorreremo, ma purtroppo nella nostra Italia si utilizzano anche tali sistemi. utilizzano anche tali sistemi. Appare, quindi, di tutta evidenza come non si possa non giudicare favorevolmente la volontà di voler mettere mano a tale importante settore con l'obiettivo di combattere quella vera e propria piaga sociale del nostro Paese costituita dalle cosiddette Tutto va bene, quindi, quando si parla di riordino e di riassetto e quando si ritiene assolutamente doveroso ed opportuno inserire all'interno di un testo unico tutta la normativa, in modo da semplificarla, razionalizzarla, renderla più intelligibile. Tuttavia, ancora una volta dobbiamo fare i conti con il metodo con il quale la maggioranza ed il Governo si rapportano con il Parlamento, come ha ricordato bene il collega Malan, ed il Paese che da questo è rappresentato. Vi è un contrasto stridente tra gli intendimenti ed il provvedimento che oggi è sotto gli occhi di questo ramo del Parlamento, che non affronta la discussione con la volontà di elaborare una legge, la migliore possibile per cercare di risolvere tale drammatica problematica, bensì si limita a delegare al Governo i successivi passaggi. Invero, appare possibile sollevare dubbi relativi alla stessa costituzionalità del disegno di legge, che riguardano in modo particolare la corretta applicazione dell'articolo 117 della Carta costituzionale, laddove stabilisce in modo inequivoco una competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di sicurezza del lavoro, interpretazione che è stata oggetto di due pareri del Consiglio di Stato in occasione dell'esame, durante la trascorsa legislatura, di un analogo provvedimento e del conseguente decreto delegato. Vi è poi il fatto che con la procedura della legge delega i tempi di concretizzazione si allungano notevolmente da oggi a quando il provvedimento medesimo potrà produrre i suoi effetti. Il rischio è di veder trascorrere altri uno o due anni mentre in Italia si vive una costante emergenza

sotto questo profilo, avrebbe avuto bisogno di altri strumenti e di altre metodologie. Lo diciamo ovviamente con spirito molto costruttivo, nella consapevolezza che tutte le parti politiche debbono contribuire al miglioramento di un testo, sul quale evidentemente avremo occasione di esprimere le nostre valutazioni. Lo stesso dicasi per l'impostazione di fondo che anima tutto il provvedimento in esame. In materia di sicurezza il vero problema è l'effettiva applicazione delle norme, che può essere realisticamente affrontato solo mettendo da parte il tradizionale atteggiamento formalistico che tanto condiziona i comportamenti sui luoghi di lavoro. Che l'approccio del disegno di legge delega all'esame sia essenzialmente formalistico e sanzionatorio lo dimostra il contenuto della lettera *f)*, riguardante la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale. Una legge delega che dovrebbe fissare solo i criteri e i princìpi si premura invece di indicare l'entità delle sanzioni incorrenti in una chiara violazione formale. Nel merito, il capitolo sanzioni presente nel disegno di legge delega è particolarmente gravoso, specialmente per le piccole e medie imprese. Combinando, infatti, il forte inasprimento delle sanzioni previste nello schema di legge delega con il già vigente appesantimento delle sanzioni introdotte in finanziaria, si ottiene un grado eccessivo di pressione repressiva. Per questo motivo avremmo preferito una tecnica legislativa più per obiettivi che per regole, attraverso normative non solo più facilmente accessibili, ma - quel che più conta - adattabili ai diversi contesti organizzativi e alle modalità oggi sempre più differenziate e articolate di lavoro. Il disegno di legge presentato dal collega Sacconi, oltre ad avere il pregio di essere un testo di legge già coordinato ed unificato con la legislazione esistente in materia, cosa che avrebbe permesso una immediata applicazione delle misure varate, affrontava tale problematica con un approccio diverso e a mio parere più convincente. Quel disegno di legge, infatti, faceva perno soprattutto sulle forme di controllo preventivo che, anzi, venivano definite forme di controllo sociale. Si arrivava, cioè, a definire un'azione di prevenzione diffusa e capillare sul territorio. La sanzione non può essere intesa come l'unico rimedio praticabile, il rischio altrimenti è quello di spingere molte piccole e medie realtà al di fuori della legge. Questo disegno di legge, di contro, così come concepito, rischia di non porre alcun rimedio alle morti bianche e agli infortuni sul lavoro, bensì - con i successivi decreti legislativi - di incrementarli, perché dove ci sono sanzioni durissime in genere c'è il sommerso e con questo tipo di norme si rischia di incoraggiare il sommerso. La modernizzazione dell'attuale assetto normativo del diritto del lavoro deve passare necessariamente attraverso importanti e funzionali interventi riformatori. Sulla capacità prevenzionale e sulla sicurezza del lavoro si misura il livello di civiltà di un Paese. Questo testo unico poteva costituire la base per istituire un sistema permanente di incentivi alle imprese, con criteri di premialità per quelle più virtuose e rispettose delle norme, invece nulla di tutto questo vi si legge. Non ci sono risorse per le politiche di professionalizzazione, non ci sono risorse per gli ispettori che dovrebbero essere chiamati a svolgere una funzione preventiva e non repressiva, vengono invece esasperati gli adempimenti formalistici contro le piccole imprese, prevedendo sanzioni che portano a misure interdittive radicali (sino al blocco dell'attività), colpendo anche i lavoratori in buona fede. Per questi motivi, non è possibile esprimere un voto favorevole a questo provvedimento, anche se siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è una necessità di riordino, ma un riordino che vada al di là di forme di repressione.

in considerazione della discussione che si sta svolgendo in queste ore, e che si ricollega a quanto accaduto in Aula nei giorni scorsi

che esiste da sempre nel nostro come in tutti i Paesi industrializzati e non, che va affrontato con massima responsabilità: è altrettanto vero che le modalità scelte dalla maggioranza nel nel preparare i provvedimenti che porta in Aula non possono che farci esprimere un parere fortemente critico,

problema del profitto, di colpa del sistema capitalista, di problema di libero mercato, di imprenditori assolutamente irresponsabili da questo punto di vista. Ricordo ai colleghi

lo stesso in quei Paesi che o non hanno avuto lo stesso sviluppo economico o peggio ancora quello sviluppo economico l'hanno avuto ma non hanno nella loro tradizione e storia l'impostazione liberale e di imprenditoria privata che fortunatamente esiste nel nostro Paese. Tant'è che oggi siamo qui a parlare di queste cose con, ad esempio, i colleghi appartenenti soprattutto alla sinistra radicale, che magari in gioventù e anche dopo hanno avuto dei miti sempre davanti agli occhi, quando proprio nei Paesi che per loro hanno rappresentato esempi giovanili e magari anche non più giovanili simili problematiche si presentano in maniera ben più grave. Pensiamo, per esempio, alla Cina, che negli ultimi anni ha avuto

si permetterebbe neanche lontanamente di non essere attento alle questioni legate alla sicurezza, perché quando si verifica un infortunio, piccolo, meno grave, grave o gravissimo è soprattutto l'impresa e l'imprenditore a subirne direttamente i danni maggiori e diretti. Quindi, nessun imprenditore porrebbe, se non la massima attenzione,

queste microimprese, dopo che la dissennata ideologia comunista sindacale degli anni Sessanta e seguenti

ci mettesse a posto la coscienza e, soprattutto, risolvesse i problemi. Non è questa la strada giusta per risolvere la questione. Intanto ricordo che in Italia sia prima sia soprattutto

non capitano perché rientrano in qualche fattispecie non prevista dalla normativa in essere. È assolutamente il contrario. La normativa copre anche più della realtà dei fatti, ma se ci sono poi imprese, e ne parleremo dopo, che queste normative non rispettano per prassi consolidata, è evidente che il peggioramento normativo, l'incremento di sanzioni, l'incremento di burocrazia legislativa, non porteranno ad alcun risultato. Arriveremo solo alla solita situazione italiana per cui chi le regole le rispetta, le rispettava già e continuerà a rispettarle, chi non le rispettava e non le rispetta, continuerà a non rispettarle anche con eventuali normative più severe.

Per ciò che abbiamo detto, l'altra questione fondamentale è quella della cultura del lavoro. Ripeto, non è questione di aggiungere qualche migliaio di righe di legge o pagine di *Gazzetta Ufficiale* su una questione che è già ampiamente coperta:

tempo, però le persone prendevano confidenza con i pericoli dei luoghi di lavoro da piccoli e crescevano con la capacità di distinguere le situazioni di pericolo da quelle della normalità

persone con un'alta scolarità, assolutamente non professionalizzante, che non trovano uno sbocco adeguato al loro titolo di studio, per cui spesso ripiegano su lavori immediatamente manuali, completamente avulsi dal tipo di preparazione che fino a quel momento hanno avuto. Oppure, come nel campo dell'edilizia, c'è una quantità enorme di cittadini extracomunitari

che non hanno la conoscenza fisica del lavoro e del pericolo: non si rendono conto, appunto, delle difficoltà quotidiane che potrebbero trovarsi ad affrontare. Allora, invece di fare leggi che si aggiungerebbero a leggi già esistenti e che non cambierebbero di una virgola la situazione,

guardano la televisione; martelliamole quotidianamente sulla necessità di comportarsi in maniera virtuosa e sicura all'interno dei luoghi di lavoro. Facciamola diventare cultura diffusa, ai ragazzi facciamo imparare a memoria qualche formazione di squadra di calcio in meno e qualche principio di sicurezza sul lavoro in più: quando saranno grandi gli servirà molto

Non c'è l'impianto che esplode (c'è stato quello dell'olio di colza, certo, e di fatto è stato l'unico caso negli ultimi due anni), non c'è il petrolchimico che si incendia, non c'è il ponte che cede perché l'ingegnere ha sbagliato il calcolo strutturale mentre era in costruzione. Gli incidenti avvengono nelle situazioni più banali e più stupide:

molti luoghi di lavoro pubblici sono stipendifici e non uffici che devono fornire un servizio alla collettività. Le persone ci sono, però otto sono in ufficio e due sulla strada. Basterebbe invertire i numeri e di colpo la quantità disponibile di persone a fare le cose che servono sarebbe immediatamente decuplicata. A proposito delle polemiche degli ultimi giorni sulla

la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro è un argomento fondamentale al quale è necessario dare ampia organicità in ragione delle preoccupazioni avvertite unanimemente

La tutela e sicurezza del lavoro è argomento che, in base all'articolo 117 della Costituzione, è riservato alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni; l'articolo 117 della al secondo comma, attribuisce alla potestà esclusiva dello Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali che su tutto il territorio nazionale devono essere salvaguardati. Di qui la necessità di garantire uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale. Inoltre, il recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro incide ampiamente sull'argomento al nostro esame e fa sì che sia necessario il riassetto della materia. La necessità di varare un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro è stata, peraltro, evidenziata nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, approvata all'unanimità nella passata legislatura. Quindi, già nella precedente legislatura - come è stato citato da alcuni colleghi che mi hanno preceduto - si era affrontato l'argomento. In ragione della complessità, dell'importanza e della delicatezza della materia, avrei, però, preferito che fosse affrontata non per delega, ma con la discussione di norme direttamente precettive. Il relatore ha riferito che alcuni articoli, in ragione dell'urgenza e anche in relazione ai lavori svolti in Commissione, sono direttamente precettivi. È un ibrido che ha una sua giustificazione, ma che, a mio parere, penso si possa migliorare nel prosieguo dei lavori, anche in ragione del contributo

Vi è un punto da cui a mio avviso bisogna partire per salvaguardare al massimo la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori. Infatti, la disciplina in atto in materia di sicurezza del lavoro si basa su un approccio con elevati livelli burocratici ed eccessivi adempimenti formali. Questa impostazione, che tra l'altro si uniforma più alle imprese di grandi dimensioni, non aderisce adeguatamente alle esigenze, ad esempio, delle piccole e medie imprese, che - lo sappiamo - caratterizzano fondamentalmente il sistema produttivo italiano, un sistema preso a modello anche da tanti Paesi all'estero. Proprio in ragione di questa caratteristica, e per rendere più efficace la sicurezza nei luoghi di lavoro, si rendono a mio avviso invece necessarie norme connotate da certezza e semplicità che sono il fondamentale elemento che costituisce il presupposto per l'applicabilità. Infatti, quando i provvedimenti, come è noto, sono troppo complessi, si creano difficoltà di applicazione e addirittura si rischia di peggiorare la situazione nel senso di non raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con le normative. Questo non significa che si possa accettare la non attenta e puntuale applicazione delle norme antinfortunistiche; si tratta però di non penalizzare chi le applica e di colpire e modificare radicalmente l'atteggiamento e il comportamento di chi sistematicamente non le applica. Quindi, unitamente alla semplificazione e razionalizzazione delle norme per la loro effettiva applicazione, è necessario prevedere ed ampliare più incisive ed efficaci misure di semplificazione e di controllo con modalità di assistenza e anche di collaborazione operativa. Sono processi, questi, anche lunghi, ma fondamentali per migliorare la situazione italiana in ordine alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro. In Italia, infatti, pur dovendo considerare la casistica con attenzione - ad esempio, il collega Amato ha fatto riferimento ad una casistica della sua Regione, che ci fa capire com'è la vera realtà di questi incidenti - si registra si registra un numero di incidenti sul lavoro più elevato rispetto ad altri Paesi dell'Unione Europea, pur avendo il nostro Paese una normativa, in ragione della comune appartenenza all'Unione Europea, simile a quella di altri Paesi europei. Allora, il formalismo, e anche un inasprimento sanzionatorio, addirittura forse anche repressivo, non è la strada fondamentale che potrà fare ottenere migliori risultati, anche se la deterrenza sanzionatoria è uno strumento ovvio. Invece, le considerazioni sul tema sanzionatorio dovrebbero indurci a considerare congiuntamente anche aspetti normativi a carattere premiale per i quali sono tra l'altro necessarie anche adeguate risorse finanziarie che io evidentemente sollecito. Del resto, adeguate risorse finanziare sono necessarie per lo svolgimento di attività di formazione e informazione, sia nelle scuole, sia per le figure imprenditoriali e anche dei lavoratori. È una strada lunga, forse anche costosa, ma alla quale una comunità deve prestare la massima attenzione e il massimo impegno. È un parametro di civiltà. Convengo sulla fondamentale utilità di predisporre percorsi formativi e informativi per i lavoratori per una crescita della coscienza, per una consapevolezza dei rischi nell'ambiente di lavoro. Sono anche d'accordo sull'opportunità di inserire nei programmi scolastici e nei percorsi formativi la materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Avevo citato le conclusioni unanimemente approvate da parte della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro: è urgente un migliore coordinamento degli interventi degli organi di vigilanza. Le morti e gli infortuni sul lavoro sono una piaga inaccettabile. Le autorevoli sottolineature e raccomandazioni ed anche il responsabile lavoro svolto dalla competente Commissione al Senato stanno a significare l'impegno di tutti. L'obiettivo, dunque, è quello di definire un testo - il più efficace - per cancellare questa piaga. Di qui la possibilità di migliorarlo in questa sede con l'apporto di tutti, ma anche la necessità di una maggiore disponibilità di risorse, di ridurre i formalismi a favore di una più accentuata efficacia, di un non utile inasprimento sanzionatorio a favore, invece, di un migliore sistema di controllo e monitoraggio sinergico tra Stato, Regioni, imprenditori, parti sociali, finalizzato alla prevenzione. Questa è l'impostazione, con l'informazione e formazione e con l'incentivazione del ravvedimento operoso, cui si deve aggiungere un virtuoso diritto di interpello, di interpello, recepito con un emendamento in Commissione e che contribuisce ad una maggiore responsabilità e ad una più corretta applicazione delle norme antinfortunistiche. È necessario, a mio avviso, come a parere di altri colleghi intervenuti prima di me, un approccio più innovativo per obiettivi condivisi e meno farraginosi, meno burocratici e senza inutili aggravamenti sanzionatori, sopratutto per le piccole e medie imprese e le medie aziende. Molti emendamenti proposti vanno in questa direzione. Si tratta, però, di cambiare, a mio modo di vedere, l'approccio complessivo del testo della delega. Ho qualche dubbio, ma mi auguro non vi siano atteggiamenti preconcetti,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, non possiamo certo nasconderci l'importanza dell'emanazione di un testo di legge come quello che ci apprestiamo a discutere. interessante stillicidio di notizie funeste, relativo alle cosiddette morti bianche, impone una svolta decisiva nelle politiche che riguardano il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza nel mondo del lavoro, dei luoghi dove si svolge, delle pratiche ivi poste in essere, di tutte quelle persone che quotidianamente si trovano a praticarlo a proprio rischio e pericolo. Sembra ormai non più differibile il momento, per il Governo, di assumersi la responsabilità dell'adozione di una serie di misure volte ad un radicale ridimensionamento di questo fenomeno, del tutto indegno di un Paese civile. Secondo i dati che proprio l'EURISPES, in un'indagine sugli infortuni sul lavoro, ha di recente evidenziato, il lavoro è in grado di uccidere come una guerra: tra il 2003 ed il 2006 sono morte sul lavoro 5.252 persone. Questo significa che ogni anno in Italia muoiono in media 1.376 persone per infortuni sul lavoro. E per questo sono urgenti azioni immediate da parte del Governo per arginare il tragico problema. Le morti bianche portano con sé gravi danni, umani e familiari, oltre al costo che l'intera comunità nazionale è chiamata a sostenere in termini economici e sociali, laddove alcuni imprenditori disonesti cercano di trarre addirittura un turpe profitto da risparmi sulle misure che invece dovrebbero essere adottate. La necessità di varare quanto prima il testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro ha potuto così evidenziare una piena convergenza di tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione. Si è quindi posto in essere un lavoro proficuo, che ha portato all'adozione di una delega, i cui princìpi, ma anche l'impianto generale, sono in parte condivisibili. Del resto, sembrava a tutti evidente che il punto di partenza della predisposizione di un simile testo unico non potesse configurarsi che in un intervento di razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente in materia. L'intero *corpus* normativo oggi in vigore porta infatti il peso di più di cinquant'anni di interventi legislativi, emanati senza alcuna soluzione di continuità e spesso rispondenti a logiche profondamente differenti tra loro. Il carattere disomogeneo dell'intera disciplina è stato anche aggravato dalla necessità di attuare le direttive comunitarie succedutesi dagli anni Ottanta fino ad oggi e dirette all'adozione di prescrizioni minime, comuni a tutti i Paesi dell'Unione, per migliorare le condizioni di lavoro. Quest'opera di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, peraltro assolutamente indispensabile, ha comportato l'ulteriore cumulo di disposizioni normative, della cui semplificazione e coordinamento oggi non si può fare più a meno. Da questo punto di vista, non si può negare che il testo della delega licenziato dalla Commissione, sebbene elaborato con scarso quanto inspiegabile senso della collegialità, cerchi, anche se a fatica, di andare nella direzione auspicata. Non convince pienamente, tuttavia, la soluzione adottata. Ci domandiamo, infatti, che senso possa avere concedere una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti, insieme alla contemporanea previsione di una serie di nuove norme. L'elaborazione di un provvedimento di delega, che si ritenga debba prevedere anche un contenuto del tutto innovativo, impone evidentemente la predisposizione di criteri direttivi chiari, completi e vincolanti per l'organo che dovrà emanare il provvedimento conclusivo. Se l'esigenza è veramente quella di semplificare e coordinare una materia intricata e complessa quale quella in oggetto, la soluzione, per così dire ibrida, che andiamo a esaminare non sembra certo quella più razionale. Una soluzione mista del tutto manichea, che, da un lato, prevede norme specifiche immediatamente vincolanti per il Governo, che sarà chiamato poi al riassetto della materia, e, dall'altro, risolve invece la successiva delega nel dare con una certa superficialità totale carta bianca al Governo. A mio avviso, siamo di fronte a un'evidente contraddizione nel momento in cui si concede al Governo una grande libertà di manovra attraverso l'indicazione di criteri del tutto vaghi e generici per il riordino della materia, salvo poi vincolarla al rispetto di alcune norme specifiche, che il Governo non si può certo permettere di smentire di qui a pochi mesi per non entrare in evidente contraddizione con la sua maggioranza. L'estrema genericità della delega, peraltro, determina il rischio che l'attività parlamentare possa perdere molta della sua efficacia emendativa, mentre espone il Governo a una deriva autocratica del tutto superflua in relazione alla materia, anche potenzialmente dannosa in questo clima di continua e reciproca delegittimazione. Forse si poteva rimandare all'Assemblea parlamentare l'esame e la definizione dell'intera materia, procedendo quindi con la più ampia partecipazione di tutte le forze politiche all'emanazione di un testo unico per quanto questo sì sarebbe stato allora un testo veramente di riassetto e riforma dell'intera normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro. Contro una simile scelta non poteva certo addursi l'argomento di una maggioranza risicata, che avrebbe reso difficile il dibattito e mortificato la decisione; anzi, vista la delicatezza della materia, proprio le difficoltà numeriche avrebbero potuto esaltare il senso di responsabilità della nostra Assemblea, fin troppo esposta a critiche di inerzia in questa legislatura. Né del resto può essere addotto il pur lodevole argomento della necessità di accelerare il processo di definizione normativa, stanti i tempi veramente lunghi che questa delega concede al Governo. In un Paese che sconta una tragica media di circa tre morti al giorno lasciare al Governo un termine di nove mesi appare al comune buon senso francamente eccessivo, soprattutto se si considera che molte delle previsioni normative contenute in questa delega saranno costrette poi a scontare una carenza di copertura finanziaria. Questo mi sembra un punto sconcertante sul quale è doveroso porre l'accento. Nonostante si abbia in cassa quello che comunemente viene chiamato un tesoretto, ci domandiamo come mai nessuno abbia realmente previsto di dedicarne una buona parte a garantire la quanto più celere possibile entrata in vigore delle norme e degli istituti previsti in questa materia. Delle due l'una: o non si è convinti della possibilità di pervenire ad un testo realmente efficace e incisivo sul problema (e allora stiamo perdendo tempo, con buona pace dei problemi del Paese che siamo chiamati a risolvere), oppure avete esigenze di cassa più pressanti, che sinceramente oggi qui in questa sede a noi sfuggono. Da un punto di vista normativo, comunque, lo stesso provvedimento non sembra sia particolarmente originale, né innovativo. Innanzitutto, il testo che ci troviamo oggi di fronte non sembra ancora in grado di cogliere la peculiarità delle piccole imprese rispetto alle medie o, addirittura, alle grandi in una materia che presenta equilibri così delicati. Trattasi di specificità di non poco conto che non hanno rilievo solo sui maggiori oneri economici, ovvero sugli aspetti sanzionatori che in entrambi i casi possono anche diventare sproporzionati, ma che possono arrivare a confliggere con il senso stesso delle norme che andiamo ad introdurre favorendone la disattenzione e la mancata applicazione. Il decreto legislativo n. 626 del 1994, che sembra tagliato su misura esclusivamente delle grandi imprese, ha finora imposto alle piccole l'enorme mole di inutili ed onerose complessità burocratiche che non trovano poi in questa delega una così pronta razionalizzazione e semplificazione, come era nei propositi. Non si tratta di fare degli sconti ad una determinata categoria produttiva piuttosto che ad un'altra, ma di realizzare un sistema che sia capace di commisurare ogni intervento non solo al criterio oggettivo del rischio, ma anche a quello soggettivo della dimensione aziendale. In questi anni di applicazione del citato decreto n. 626 è emerso chiaramente che né gli eccessi burocratici, né quelli sanzionatori possono contribuire a proteggere i lavoratori. Per garantire migliori condizioni di sicurezza bisogna, invece, puntare sulla semplicità degli adempimenti cartacei e sulla razionalizzazione del sistema dei controlli e delle sanzioni sviluppando la prevenzione e incentivando la formazione di imprenditori e dipendenti. Non può sfuggire, infatti, come l'impostazione complessiva della materia sembri ancora incentrata principalmente sul mero rispetto di regole formali e sull'erogazione delle connesse sanzioni. Queste ultime, va detto per inciso, appaiono sproporzionate e inidonee a consentire una maggiore effettività delle norme antinfortunistiche. La storia giuridica del nostro Paese avrebbe dovuto ormai insegnarci che ogni sanzione sproporzionata rispetto alla corrispondente ipotesi di reato si dimostra del tutto inadeguata a favorirne la deterrenza. Insistere su un approccio simile non significa, forse, continuare a pagare il dazio di una deriva ideologica, quanto non del tutto emotiva, che fa della sanzione l'unico strumento a disposizione per pretendere di risolvere il problema? Le ormai tristemente famose morti bianche costituiscono una piaga sociale da risolvere intervenendo alle radici del fenomeno, che sono culturali prima ancora che giuridiche. La complessità del tema e l'importanza dei valori in gioco impongono, infatti, la promozione di un vero e proprio cambiamento di passo. Si sente il bisogno che il maggiore rispetto della normativa vigente si possa fondare non solo sul consueto meccanismo sanzionatorio (la cui effettività, peraltro, risente di una cronica mancanza di risorse e mezzi), ma anche sulla predisposizione di un percorso che sia capace di venire incontro alle carenze di formazione, informazione e prevenzione. Il cambiamento dell'atteggiamento culturale è uno strumento di gran lunga più efficace di ogni meccanismo sanzionatorio e da questa delega sembrava doveroso aspettarsi un'inversione di tendenza che, allo stato attuale, ancora non c'è stata. In Commissione abbiamo più volte perorato la causa di un percorso di formazione preventiva che insegni le indispensabili misure di sicurezza ai lavoratori e agli imprenditori, soprattutto ai più giovani, inesperti e, per questo, maggiormente esposti e questo già a partire dall'insegnamento scolastico. Abbiamo poi insistito anche sulla predisposizione urgente di mezzi e risorse per una maggiore collegialità degli organi preposti alla prevenzione e al controllo di una migliore efficienza della loro attività. La formazione preventiva ed un efficace coordinamento ispettivo sono i primi passi di una realistica inversione di tendenza. Ma per fare questo occorre che vengano immediatamente destinate allo scopo risorse aggiuntive, anche consistenti, senza le quali il Governo rischia di predicare bene e a razzolare male ad un prezzo, questa volta, che non possiamo proprio permetterci di pagare. Il senso di responsabilità nei confronti del tema, particolarmente tragico, cui peraltro lo stesso Presidente della Repubblica ci ha più volte richiamati, ci impone di non abbandonare un testo che fin qui, per tutto quello che è stato detto, non sembra condivisibile. Auspichiamo pertanto che il dibattito nelle Aule parlamentari possa introdurre significativi miglioramenti nelle direzioni indicate.

Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che oggi ci troviamo ad esaminare reca misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo il riassetto e la riforma della normativa in materia. Anzitutto, va osservato che questa è una materia di fondamentale importanza, considerato il grande e doloroso tributo di vite umane e di conseguenze negative sulla salute dei lavoratori che ogni anno si paga in materia di infortuni sul lavoro. Con questo provvedimento il Parlamento viene completamente esautorato e l'opposizione privata della elementare nonché costituzionalmente garantita possibilità di dire la sua in questa delicata materia. Tutto ciò per il solito motivo che ormai è diventato il tormentone di questa legislatura e che riguarda tutti i provvedimenti di un certo rilievo, e cioè l'assoluta mancanza di posizioni univoche da parte di questa maggioranza e di questo Governo sui temi di maggiore importanza per il Paese ed il terrore di andare sotto, vista la maggioranza risicata di numeri soprattutto al Senato. Viene comunque spontaneo chiedersi quali siano le cause di tutti questi incidenti sul lavoro e le risposte possono essere sostanzialmente due: non esiste una normativa idonea ad arginare e contrastare efficacemente il fenomeno; esiste una normativa compatibile con le esigenze di salvaguardia della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro, ma queste norme non vengono applicate. Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè quello della normativa vigente in materia, vanno sicuramente menzionati il decreto legislativo n. 626, recante normativa sulla sicurezza del lavoro e, in materia di sicurezza antincendio, il decreto n. 139. Questa normativa (in particolare il decreto legislativo n. 626) risulta essere fortemente incisiva e pone le condizioni necessarie affinché sui luoghi di lavoro siano osservati determinati comportamenti minimi posti a tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Semmai, questa normativa necessiterebbe di una rivisitazione e della riunione di tutte le norme in un Testo unico. Quindi se è vero come è vero che la normativa attuale, con una parziale rivisitazione, è già sufficiente a svolgere quell'opera di prevenzione alla quale è preposta, vuol dire che questa non viene attuata e che in particolare non vengono effettuati i controlli dagli organismi a questo compito demandati. Molto spesso, quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, si pensa al settore della cantieristica ed in particolare dell'edilizia, mentre forse non si ha il coraggio di dire che, in base al ricordato decreto legislativo n. 626, se oggi fossero effettuati dei controlli rigorosi, ci troveremmo ad assistere alla chiusura di buona parte degli uffici pubblici, delle scuole, degli ospedali, dei Ministeri e via dicendo. Quindi il problema, signor Presidente, non sta nel colmare un vuoto legislativo inesistente, ma nell'effettuazione di controlli capillari sul territorio da parte delle autorità a ciò preposte. Allora, ci dobbiamo chiedere quale sia la logica che sottostà all'adozione di un provvedimento come quello che oggi ci troviamo di fronte. La logica - ahimè è sempre la stessa ed è quella di gravare le imprese di inutili adempimenti per coprire le manchevolezze dell'apparato dello Stato, che non effettua adeguati controlli. legislativo n. 626 impone alle imprese un'attività tale da comportare dei costi elevatissimi, sia per i lavori da effettuare che per le unità di personale da impiegare nelle verifiche periodiche. Ma tutti questi discorsi questo Governo e la sua maggioranza hanno un approccio culturale sbagliato, salvo poi meravigliarsi quando nelle aree economicamente più progredite del Paese si perdono le elezioni con percentuali bulgare, come accaduto di recente nell'ultima tornata tornata di elezioni amministrative. Non riflettete a sufficienza sul fatto incontestabile che le imprese, ed in particolare quelle di dimensioni medie e piccole, costituiscono il volano dell'economia di questo Paese e che le classi produttive dello stesso sono stufe di dover combattere quotidianamente, da un lato, la lotta derivante dalla concorrenza dei mercati esteri e, dall'altro, quella contro le inutili vessazioni proposte da questo Governo e figlie di un retaggio ideologico che ormai dovrebbe essere morto e sepolto. Un altro fronte sul quale il Governo attuale e la maggioranza che lo sostiene dovrebbero abbondantemente riflettere è quello del lavoro nero, privo di qualunque minima garanzia per i lavoratori e quasi sempre dovuto all'inerzia nel settore dei controlli del personale preposto alla vigilanza contro il verificarsi del fenomeno. Non si riesce a capire il perché in determinate zone del Paese (situate prevalentemente nel Mezzogiorno), l'impiego irregolare di manodopera costituisca di fatto, la norma, un personale, come ricordato, senza alcuna tutela, mal pagato ed esposto a tutti i rischi ivi compresi quelli legati alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Ma anche di questo nessuna traccia, non si legge da nessuna parte neanche la mera intenzione di questo Governo in carica e della sua maggioranza di stanziare i fondi necessari per l'effettuazione dei necessari controlli da parte degli organismi a ciò deputati. La volontà punitiva di questo Governo e della sua maggioranza nei confronti delle imprese e quindi della classe produttiva del Paese, emerge in modo chiaro dall'analisi del sistema sanzionatorio contenuto Questo risulta fortemente sproporzionato se rapportato a quello applicato alla commissione di altre fattispecie criminose di uguale rilevanza. Punire, quindi, senza rendere efficiente il sistema. Teniamo presente inoltre che non solo un innalzamento del sistema dei controlli potrebbe autofinanziarsi attraverso i proventi che deriverebbero dall'emersione del lavoro nero, ma con ogni buona probabilità deriverebbero da questo una massa di risorse tali da poter essere destinate ad altri bisogni dei lavoratori. Un altro aspetto inquietante è che tutto questo dibattito si svolge contemporaneamente ad un altro disegno di legge, che è stato all'esame del Senato in questi giorni, che è rubricato «Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio dello Stato». Senza entrare nel merito di tale provvedimento e dell'incongruenza di chi, da un lato, vorrebbe agevolare l'ingresso di clandestini nel nostro Paese e, dall'altro, si propone di contrastare lo sfruttamento degli stessi, si deve purtroppo notare che questo scellerato Governo ha maggiormente a cuore la salvaguardia dei cittadini stranieri entrati illegalmente in questo Paese anziché la maggior parte dei giovani e meno giovani del Sud che, come già ricordato, svolgono lavori precari, privi di ogni tutela e carenti dal punto di vista della sicurezza dei luoghi di lavoro. Pertanto, signor Presidente, la soluzione seria di questa problematica, che ci porterà, se attuata puntualmente, ad un drastico calo di infortuni sul lavoro e delle conseguenze a questi legate, passa inevitabilmente attraverso la piena applicazione di quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 626 opportunamente rivisitato. l'intensificazione dei controlli da parte delle autorità preposte al rispetto della normativa vigente: controlli diffusi sui luoghi di lavoro pubblici e privati e controlli a tappeto per favorire l'emersione del lavoro nero e contro la situazione di sfruttamento in cui vivono molti dei nostri giovani. Signor rappresentante del Governo, colleghi della maggioranza, abbiate per una volta il coraggio di smetterla con le mistificazioni ed inquadrate realmente i problemi e le loro soluzioni concrete, abbandonando questo inutile provvedimento e destiniamo le risorse necessarie all'effettuazione dei controlli da parte degli organismi pubblici a ciò deputati. Del resto, le risorse per finanziarie la fase iniziale ci sono: avete il "tesoretto" realizzato grazie al buon governo del Paese nei cinque anni dell'Esecutivo Berlusconi, che con una riduzione della tassazione ha dato modo a tutti di pagare le tasse; così si è formato l'extragettito, sull'impiego del quale ogni giorno sentiamo proporre da voi ogni sorta di possibile destinazione, molto spesso anche in contrasto con gli interessi reali del Paese. Investiamo quindi nell'intensificazione dei controlli e nella vera salvaguardia dei lavoratori e restituiamo loro, sotto forma di maggiori garanzie, una parte di quanto gli è stato sottratto attraverso il prelievo fiscale. Per quanto esposto, la nostra valutazione su questo provvedimento è fortemente negativa.

Presidente, sto per presentare un'interrogazione al Ministro del lavoro, perché credo che oggi sia avvenuto un fatto grave: Confcooperative è stata esclusa dalla composizione del rinnovato consiglio d'amministrazione dell'ENASARCO,